L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che in data 30 novembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2031). finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19».

è trascorso meno di un mese da quando, il 6 novembre, con la mia ultima informativa ho riferito al Parlamento sull'evoluzione della pandemia in Italia e sulla prima ordinanza da me firmata il 4 novembre in attuazione del DPCM del 3 novembre. Adesso, con il rispetto che si deve al lavoro del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, seguirò attentamente le osservazioni, le proposte e gli indirizzi che verranno formulati nel corso di questo dibattito parlamentare da tutte le forze politiche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. La seduta odierna assume un'ulteriore rilevanza perché nella seconda parte del mio intervento intendo illustrare le linee guida del nostro piano strategico sui vaccini COVID, elaborato dal Ministero della salute, dal Commissario straordinario per l'emergenza, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale Nei principali Paesi europei un passaggio parlamentare come questo non è ancora avvenuto. Io penso che sia fondamentale il pieno coinvolgimento del Parlamento su una sfida così strategica per il futuro del Paese. Consiglio dei ministri e naturalmente dal quadro epidemiologico da cui esso deriva. Prima di soffermarmi sugli effetti che hanno avuto le ordinanze firmate in queste quattro settimane, mi preme ricordare che il Governo, già prima del DPCM del 3 novembre, dinanzi all'aumento del numero dei contagi e dell'indice RT, aveva assunto misure più stringenti per contrastare una diffusione incontrollata dell'epidemia. Le mie ordinanze sono state adottate, come prescritto dalla norma, sulla base della classificazione delle Regioni, effettuata con cadenza settimanale dalla cabina di monitoraggio, sentiti i Presidenti di Regione e il nostro comitato tecnico-scientifico. Sono scelte dettate da valutazioni scientifiche, ispirate come sempre al principio di precauzione, e dalla nostra ferma volontà di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, come indica la nostra Costituzione. Sono scelte che, come dimostrano gli ultimi dati, hanno aiutato le Regioni prima a rallentare l'espansione del contagio e poi a ridurre, anche in valore assoluto, il numero quotidiano dei nuovi casi. Il Governo, attraverso le mie ordinanze, si è assunto la responsabilità di scelte difficili quanto necessarie. Ogni ordinanza restrittiva comporta sacrifici di cui siamo ben consapevoli, ma senza queste scelte sarebbe impossibile mettere la curva sotto controllo. La pressione sulle strutture ospedaliere diverrebbe insostenibile: non reggerebbero i nostri medici, gli infermieri e tutti i professionisti sanitari, cui va sempre la nostra più convinta gratitudine per il lavoro incessante che stanno svolgendo. *(Applausi)*. I dati dell'ultima rilevazione della cabina di monitoraggio e, in modo particolare, il lavoro incessante dell'Istituto superiore di sanità ci forniscono indicazioni certamente molto utili per orientare le nostre prossime scelte. Dall'analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l'insieme delle misure che abbiamo adottato inizia a dare i primi incoraggianti risultati: diminuisce l'incremento quotidiano dei contagi e tutto lascia prevedere che la prossima rilevazione del monitoraggio dovrebbe confermare la tendenza in discesa dell'indice RT, che è passato in quattro settimane da 1,7 a 1,4, a 1,2, a 1,08. Sono fiducioso che a breve l'indice possa scendere sotto l'1 e questo, come è noto, è un elemento essenziale per riportare il contagio sotto controllo. La situazione è molto seria in tutto il Paese e nessuna sottovalutazione può essere ammissibile, però mi sembra giusto sottolineare dinanzi al Parlamento quella che è una verità ormai evidente: le misure che abbiamo messo in campo come Governo e come Regioni stanno funzionando e le valutazioni dei nostri scienziati si stanno rilevando fondate. A marzo fu l'Italia, con coraggio e determinazione, ad indicare agli altri Paesi occidentali la strada del *lockdown* per fermare la pandemia; adesso, nella seconda ondata, stiamo sperimentando una strada diversa. L'obiettivo del Governo è piegare la curva senza un *lockdown* generalizzato, che invece altri Paesi sono stati costretti a scegliere. L'esperienza di queste settimane ci dice che la nostra scelta di adottare un modello per classificare le Regioni in base allo scenario e al livello di rischio e di modulare proporzionalmente le misure da adottare appare in grado di appiattire la curva del contagio, senza ricorrere nuovamente a un *lockdown* totale in tutto il Paese, con i costi sociali ed economici che esso comporterebbe. È un risultato non scontato, sul quale non mi soffermo oltre, perché oggi mi preme parlare innanzitutto di quel che dobbiamo fare domani e nelle prossime settimane, più che rivendicare i primi passi avanti fatti. Io credo che sia indispensabile avere gli occhi bene aperti. Guardare i progressi che stiamo compiendo grazie alle misure adottate non può significare non vedere, con altrettanta nitidezza, le grandi difficoltà che permangono. I dati evidenziati dall'ultima rilevazione della cabina di monitoraggio sono molto chiari: guai a non leggerli tutti con la stessa attenzione. Siamo in presenza di una sostenuta circolazione del virus, che rende molto difficile il *contact tracing* e può alimentare nuovi consistenti focolai e siamo in presenza di una forte pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive e sull'area medica. Per la stabilizzazione dei primi risultati positivi di cui ho parlato, c'è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una robusta cura di mantenimento. Lo dico con tutta la forza che ho dentro: attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo, l'onda resta ancora molto alta e la nostra navigazione continuerà ad essere difficile ed esposta a mille imprevisti, lo dico con la chiarezza e la forza che deve avere in questi passaggi il Ministro della salute. Non facciamoci illusioni: se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l'angolo. Ripeto ancora una volta un'espressione che ho usato mille volte in questi mesi: non dobbiamo perdere la memoria, conosciamo ormai il virus, sappiamo i danni che fa e la facilità con cui se ne può perdere il controllo. In troppi, nei mesi susseguenti al *lockdown*, hanno frettolosamente teorizzato che il virus avesse perso forza, che il rischio di una seconda ondata era sostanzialmente inesistente, che si poteva fare a meno dell'obbligo di rispettare le regole, a partire dall'utilizzo delle mascherine. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si è pericolosamente abbassata la soglia di attenzione e il rispetto delle tre regole fondamentali di prevenzione (mascherine, distanziamento, igiene delle mani) e si è determinato un clima da liberi tutti sbagliato e ingiustificabile. Ricordo questi fatti con preoccupazione, senza voler alimentare polemiche che non servirebbero a nulla, unicamente per rinnovare un monito ed un allarme che ho ripetuto più volte anche dopo il *lockdown* e prima dei mesi estivi. Voglio ricordare alcuni numeri che dobbiamo avere sempre ben impressi, perché non si ripetano nelle festività natalizie le stesse leggerezze viste in estate. Il 20 marzo, nella giornata più drammatica della prima ondata, abbiamo registrato 6.237 casi, dopo il *lockdown* a luglio la media giornaliera era scesa a 237 casi al giorno, ad agosto eravamo a 778, a settembre la media è salita a 1.608, con una punta massima di 2.588 casi. Nel mese di settembre - questo è il punto il virus ha iniziato a rompere gli argini, a tracimare, uscendo dai confini dentro i quali eravamo riusciti a tenerlo. Ammesso che qualcuno coltivi ancora dubbi sulla forza e sulla velocità di propagazione del Covid, voglio ricordare brevemente ancora qualche altro dato. Nella settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre abbiamo avuto 14.587 casi, in quella successiva 28.196, poi 52.960, poi 100.446, poi 183.243, poco meno di un raddoppio settimanale. Nella settimana che va dal 2 all'8 novembre, è iniziato leggermente a diminuire l'incremento, con 200.829 casi, che sono divenuti poi 211.850 in quella successiva. Nell'ultima rilevazione della cabina di monitoraggio c'è la prima riduzione in valore assoluto del numero dei contagi, che sia assesta a 193.309, con una media di 27.615 al giorno ed un indice Rt, come dicevo, pari a 1,08. Dal rilevamento di fine settembre-inizio ottobre alla settimana scorsa, il tasso medio di occupazione dei posti letto in area medica è passato dal 7 per cento a circa il 50 per cento e quello delle terapie intensive dal 4 per Questi numeri non credo abbiano bisogno di particolari commenti. A settembre, dopo il *lockdown*, eravamo mediamente a 1.608 casi al giorno, adesso abbiamo dati certamente in diminuzione, ma siamo ancora ieri sera a 19.350 nuovi contagi, il picco più alto delle ultime settimane era stato sopra i 40.000 casi. del tutto evidente che con tale circolazione del virus, se abbassiamo la guardia, andiamo incontro a un esito segnato. Abbiamo un'incidenza di 320 casi circa ogni 100.000 abitanti. Dobbiamo arrivare a 50 casi ogni 100.000 abitanti. ragione le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà, se non vogliamo nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio. Ripeto ancora una volta un concetto per me basilare: senza consistenti limitazioni dei movimenti, un cambio sostanziale delle nostre abitudini e un rigoroso rispetto delle regole di sicurezza, la convivenza con il virus fino al vaccino è destinata al fallimento. Questa è la verità che è dinanzi a noi. In società fortemente sviluppate come la nostra, senza ridurre gli spostamenti e le occasioni di contagio, la convivenza con il virus è difficilmente realizzabile. Per questo con il prossimo DPCM dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose, anche per non vanificare il lavoro fatto nelle ultime settimane. Gli orientamenti del Governo possono essere riassunti in due scelte di fondo. di riconfermare il modello della classificazione delle Regioni per scenario e indice di rischio. Il sistema delle tre zone (rossa, arancione e gialla) ha dato risultati che riteniamo soddisfacenti. I tecnici del Ministero, assieme a quelli dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni, si stanno confrontando sui parametri, ma l'impianto di fondo è corretto e sta funzionando. È uno strumento efficace che ci consente di agire rapidamente e in modo proporzionale al variare delle condizioni epidemiologiche. Oggi, in un contesto di primo miglioramento, le Regioni tendono verso il giallo, ma qualora il quadro dovesse peggiorare abbiamo già vigente uno strumento automatico che può subito riattivare misure più restrittive. seconda scelta. Per affrontare adeguatamente le festività natalizie e quelle di fine anno le limitazioni previste dovranno essere rafforzate, anche nel quadro di un coordinamento europeo che il nostro Paese ha promosso nelle ultime settimane. Tale coordinamento è sempre utile - questo è il mio punto di vista ma diventa indispensabile se si pensa ad attività che si svolgono sui confini naturali tra Stati diversi. In questo contesto appare necessario limitare il più possibile i contatti non indispensabili tra le persone. L'orientamento del Governo - e su questo ascolterò con attenzione gli indirizzi delle Camere - è che durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali e limitati gli spostamenti tra le Regioni, come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni. Inoltre, nei più importanti giorni di festa - il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio - vanno limitati anche gli spostamenti tra i Comuni. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. È opportuno, più in generale, ridurre i rischi di diffusione del contagio connessi ai momenti di aggregazione durante le festività del Natale e del Capodanno. Si tratta di misure indispensabili se non vogliamo vanificare i primi segnali di miglioramento. Non sarà un Natale come gli altri, ma serve davvero il contributo di tutti per ridurre il numero dei contagi quello, purtroppo molto alto, dei decessi, nonché per alleggerire la pressione sulle nostre strutture sanitarie. Abbiamo scelto consapevolmente di mantenere le lezioni in presenza nella scuola primaria e nella prima media anche nelle zone rosse. È una scelta che rivendichiamo e che si connette con la centralità che le attività scolastiche assumono nella vita delle nostre comunità. Con l'uscita di molte Regioni dalle zone rosse è già in corso anche una ripresa delle lezioni in presenza per le classi di seconda e terza media. Compatibilmente con l'evoluzione del quadro epidemiologico, è obiettivo del Governo riportare gradualmente in presenza anche gli studenti delle scuole superiori. Vengo ora alla seconda parte del mio intervento, relativa al piano strategico dei vaccini Covid. Intendo, in via preliminare, svolgere due considerazioni che ritengo molto importanti e decisive. Innanzitutto, dopo le parole crude che ho utilizzato per sottolineare i tanti rischi che sono ancora dinanzi a noi, mi preme evidenziare con la stessa nettezza un chiaro messaggio di speranza. Dopo mesi difficilissimi e giornate che non dimenticheremo mai, il messaggio di fondo che voglio rivolgere al Parlamento e, attraverso di voi, a tutti gli italiani, è un messaggio di ragionata fiducia. Cari colleghi, dentro la tempesta che ancora stiamo vivendo, finalmente vediamo un approdo, abbiamo una rotta chiara verso un porto sicuro. Adesso è possibile perché appare probabile che, a partire da gennaio, avremo i primi vaccini e poi, progressivamente, saremo in grado di vaccinare un numero sempre più alto di italiani. È la svolta che auspichiamo e alla quale lavoriamo da mesi; siamo stati i primi in Europa, assieme a Germania, Francia e Olanda, a costruire l'alleanza per i vaccini nel mese di maggio e a porre il tema di un impegno comunitario perché si investisse sulla ricerca e su tutte le sperimentazioni. Ora, finalmente, vediamo i primi risultati. Serve ancora prudenza e serve ancora cautela. La verità è che al momento, mentre vi parlo, nessun vaccino è stato approvato né dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), né dall'agenzia statunitense I segnali che arrivano però dagli studi effettuati sono incoraggianti e ci hanno portato ad accelerare la definizione del piano strategico che individua le linee essenziali di visione ed azione che intendiamo adottare. Dal piano strategico che illustro oggi in Parlamento deriverà poi un piano esecutivo che sarà adeguato permanentemente sulla base dei processi autorizzativi delle agenzie regolatorie e della conseguente, effettiva disponibilità dei vaccini. Ho sempre pensato che la scienza ci avrebbe portato fuori da questa crisi. Ancora è presto e - lo ribadisco - serve cautela, ma si vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Al momento non è intenzione del Governo disporre l'obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna valuteremo il tasso di adesione dei cittadini. Il nostro obiettivo è senza dubbio raggiungere al più presto l'immunità di gregge. Oggi più che mai serve il contributo di tutti, con comportamenti responsabili per affrontare questa fase di transizione e di resistenza. Sono sacrifici con una scadenza temporale definita, che ci porteranno finalmente a chiudere questa pagina difficile della storia del nostro Paese, dell'Europa e dell'intera umanità. Dobbiamo compiere ogni sforzo per non far coincidere la campagna di vaccinazione con una nuova fase di grave diffusione del Covid. La campagna di vaccinazione sarà imponente e richiederà uno sforzo senza precedenti. Dobbiamo evitare di arrivarci con i nostri presidi sanitari in difficoltà e con il personale totalmente impegnato nella lotta contro il Covid. La seconda considerazione che voglio svolgere è relativa al clima politico con il quale affronteremo la stagione di vaccinazione Covid. La piena riuscita della campagna di vaccinazione deve rappresentare un obiettivo fondamentale di tutto il Paese. Non ci può essere su questo tema alcuna divisione tra noi, non possiamo permettercelo; su questo tema e su questa sfida serve un grande patto Paese con tutti dentro, nessuno escluso, non c'è maggioranza ed opposizione, ma gli italiani e il loro fondamentale diritto alla salute come precondizione indispensabile per una solida ripresa economica. È partendo da queste considerazioni di carattere generale che voglio, entrando nel dettaglio, illustrare al Parlamento le linee fondamentali del piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19). Il primo asse è tanto semplice quanto importante: l'acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. *(Applausi)*. Il vaccino è un bene comune, un diritto che va assicurato a tutte le persone, alle donne e agli uomini, indipendentemente dal reddito e dal territorio nel quale ciascuno vive o lavora; nessuna diseguaglianza sarà ammissibile nella campagna di vaccinazione. Il secondo asse è altrettanto importante e rende concreto il principio precedentemente annunciato. L'Italia ha opzionato 202.573.000 dosi di vaccino, che rappresenterebbero una dotazione sufficientemente ampia per poter potenzialmente vaccinare tutta la popolazione e conservare delle scorte di sicurezza. Con le conoscenze oggi a nostra disposizione è molto probabile che saranno necessarie due dosi per ciascuna vaccinazione, a breve distanza temporale. Va inoltre ricordato che non vi è ancora evidenza scientifica sui tempi esatti di durata dell'immunità prodotta dal vaccino. La scelta compiuta anche in questo caso è ispirata al principio di massima precauzione. Abbiamo sottoscritto, infatti, in quota parte, per la parte che riguarda l'Italia, pari al 13,46 per cento, tutti i contratti che l'Unione europea ha formalizzato. Non vogliamo correre neanche il più piccolo rischio di non poter disporre di un vaccino autorizzato prima di altri o che dovesse risultare più efficace, in conseguenza della scelta di non partecipare ad una delle acquisizioni stipulate dall'Unione europea. Non abbiamo mai esercitato il diritto di *opting-out* che era previsto dagli accordi europei. Vorrei ancora ricordare che questo meccanismo europeo di acquisto dei vaccini è stato promosso e favorito da un'iniziativa dell'Italia. Infatti, dalla prima intesa per la fornitura dei vaccini siglata il 13 giugno tra Italia, Germania, Francia e Olanda è poi scaturita la decisione dell'Unione europea di centralizzare a Bruxelles la negoziazione e la stipula di tutti i contratti. Non sono dunque i singoli Stati a trattare con le case farmaceutiche, ma è la Commissione a negoziare per conto di tutti i Paesi europei. La Commissione europea e gli Stati membri hanno infatti sottoscritto un accordo in base al quale i negoziati con le aziende produttrici sono stati affidati in esclusiva alla stessa Commissione, affiancata da un gruppo di sette negoziatori in rappresentanza degli Stati membri (tra i sette è rappresentata l'Italia) e da uno *steering board,* che assume le decisioni finali, ove siedono rappresentanti di tutti gli Stati membri. Le trattative avviate si sono concentrate su un gruppo di aziende che stanno sviluppando vaccini con diversa tecnologia. Queste dosi saranno distribuite agli Stati membri - come dicevo - in proporzione alle rispettive popolazioni a partire dal primo trimestre del 2021 e con una più significativa distribuzione delle dosi nel secondo e nel terzo trimestre, per completarsi sostanzialmente nel quarto trimestre del prossimo anno. Se tutti i processi autorizzativi andassero a buon fine - cosa su cui non possiamo, per le ragioni che prima dicevo, ancora avere certezza assoluta - l'Italia potrebbe contare sulla disponibilità delle seguenti dosi: contratto con AstraZeneca 40,38 milioni di dosi, per il contratto con Johnson & Johnson 26,92 milioni di dosi, per il contratto con Sanofi 40,38 milioni di dosi, contratto con Pfeizer-BioNTech 26,92 milioni di dosi, per il contratto con CureVac 30,285 milioni di dosi, contratto con Moderna 10,768 milioni di dosi. Sono chiaramente numeri ancora subordinati a processi autorizzativi che non sono ancora completati. Il terzo asse tempo relativo all'autorizzazione dei vaccini che abbiamo acquistato. A tal proposito, voglio innanzitutto sottolineare che la corsa contro il tempo che la comunità scientifica sta compiendo cammina di pari passo con la massima sicurezza e il pieno rispetto di tutti i protocolli di garanzia e di controllo. Disporre di vaccini efficaci e sicuri è una priorità che non può essere subordinata o condizionata da qualsiasi altro interesse. Attorno a questo impegno si determina anche un'importante responsabilità sociale d'impresa. Voglio essere chiaro: la produzione e la distribuzione del vaccino non può essere regolata unicamente dalle leggi del mercato. Su questo ho trovato molto efficace il parere inviatomi dal professor Lorenzo D'Avack, presidente del Comitato nazionale per la bioetica, che voglio ringraziare per la disponibilità e per il prezioso contributo dato. Si legge in quel parere che l'emergenza non deve portare a ridurre i tempi o addirittura ad omettere le fasi della sperimentazione, definite dalla comunità scientifica internazionale, requisiti indispensabili sul piano scientifico, bioetico e biogiuridico per garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di un farmaco. L'Europa ha scelto questa strada, non abbreviando le fasi di studio e sperimentazione dei candidati vaccini e continuando a subordinare la messa in commercio al parere definitivo e vincolante dell'EMA. L'accelerazione dei tempi è stata realizzata facendo procedere in parallelo le diverse fasi di sperimentazione, produzione ed autorizzazione. Infatti, parallelamente agli studi preclinici e clinici di fase uno, due e tre, si è avviata la preparazione della produzione su scala industriale ai fini della distribuzione commerciale. Contestualmente, l'Agenzia europea per i medicinali, l'EMA, onde contribuire all'accelerazione del processo, senza venir meno al proprio fondamentale ruolo, sta procedendo con una procedura finalizzata definita di *rolling review*, che consiste nel valutare le singole parti del *dossier* mano a mano che vengono presentati dalle aziende, anziché attendere l'invio di un *dossier* completo. Tale procedura, senza inficiare la valutazione complessiva, abbrevia significativamente i tempi e può creare le condizioni perché si arrivi a concedere una prima autorizzazione all'immissione in commercio già entro l'anno. Ad oggi sono state indicate due date da EMA, che potrebbe esprimersi il 29 dicembre sul vaccino Pfizer-Biontech e il 12 gennaio sul vaccino Moderna. Queste due aziende nel primo trimestre dell'anno prossimo da contratto dovrebbero fornirci rispettivamente 8,749 milioni di dosi Pfizer-Biontech e 1.346.000 di dosi Moderna. Mentre vi parlo non ci sono altre date fissate da EMA. Voglio ricordare che i contratti sottoscritti dalla Commissione europea, da cui discendono le distribuzioni al nostro Paese, vanno sempre considerati come *best scenario* e sono ovviamente subordinati ai processi autorizzativi che - ribadisco - non hanno ancora certezza assoluta. Noi dobbiamo essere pronti allo scenario migliore e poi adattarci se le scadenze dovessero cambiare a causa del dilungarsi dei processi di autorizzazione delle agenzie regolatorie. Il cuore della campagna vaccinale, secondo i dati di cui disponiamo e secondo le nostre previsioni, sarà comunque l'arco di tempo tra la prossima primavera e l'estate. Il quarto asse è relativo alle scelte delle prime categorie che dovremo decidere di vaccinare, a partire da quando arriveranno in Italia le prime dosi di vaccino. Si tratta di una scelta non facile; dobbiamo farla in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali ed europee e informando puntualmente i cittadini. Attualmente, l'Italia, come è noto, si trova nella fase di trasmissione sostenuta in comunità. In tale situazione epidemiologica, la strategia di sanità pubblica dovrà focalizzarsi inizialmente sulla diluizione diretta della morbilità e della mortalità nonché sul mantenimento dei servizi essenziali più critici. Al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali. gli operatori sanitari e socio-sanitari. Lavorando e operando in prima linea, essi hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione da Covid-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. Difendere questi professionisti in prima linea aiuterà a mantenere la resilienza del Servizio sanitario nazionale. categoria: residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Un'elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali è stata gravemente colpita dal Covid-19; i residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave a causa dell'età avanzata, la presenza di molteplici comorbilità e la necessità di assistenza per alimentarsi e per altre attività quotidiane. Pertanto, sia la popolazione istituzionalizzata sia il personale dei presidi residenziali per anziani devono essere considerati ad elevata priorità per la vaccinazione. persone in età avanzata. Un programma vaccinale basato sull'età è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore copertura vaccinale. È anche evidente che un programma basato sull'età aumenti la copertura anche nelle persone con fattori di rischio, visto che la prevalenza di comorbilità aumenta con l'età. Questo gruppo di popolazione rappresenta, quindi, un'altra priorità assoluta per la vaccinazione. Ecco alcuni numeri delle categorie sopra indicate, costruiti nel confronto con le Regioni, con Istat e con i *database* del Ministero della salute. Operatori e lavoratori sanitari e socio-sanitari: 1.404.037 persone; personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani 570.287 persone;

popolazione con almeno una comorbilità cronica: 7.403.578. Alcune di queste categorie naturalmente saranno le prime a ricevere il vaccino. Naturalmente, con l'aumento delle dosi si inizieranno a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali quali anzitutto gli insegnanti e il personale scolastico, le Forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Nel caso in cui, si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, saranno destinate eventuali scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo reattivo rispetto a quel territorio in difficoltà. Il quinto asse è relativo a logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, che saranno di competenza del commissario straordinario. Nella definizione dei piani di fattibilità e delle forniture di tutte le attrezzature, strumenti e materiali necessari, sono stati considerati diversi aspetti, tra cui la catena del freddo estrema per la conservazione di alcuni vaccini o la catena del freddo *standard*, il confezionamento dei vaccini multidose e la necessità di diluizione. Per i vaccini che necessitano di catena del freddo *standard*, compresa tra i due e gli otto gradi, si adotterà un modello di distribuzione *hub and spoke*, con un sito nazionale di stoccaggio e una serie di siti territoriali di secondo livello. Per quanto riguarda invece i vaccini che necessitano di catena del freddo estrema, questi verranno consegnati direttamente dall'azienda produttrice presso 300 punti vaccinali, che sono già stati condivisi con le Regioni e le Province autonome. Il confezionamento dei vaccini multidose richiede l'acquisto di un adeguato numero di siringhe, aghi e diluente, che è assicurato sia tramite *joint procurement* europeo, sia attraverso richiesta di offerta pubblica, già emessa dagli uffici del Commissario per l'emergenza. Il Commissario straordinario assicurerà anche il materiale ritenuto essenziale per lo svolgimento delle sedute vaccinali, a partire dai dispositivi di protezione. La distribuzione dei vaccini, in particolare di quelli relativi alla catena del freddo *standard*, avverrà con il coinvolgimento delle Forze armate, che in accordo con il Commissario straordinario stanno già pianificando vettori, modalità e logistica. Voglio a tal proposito ringraziare il ministro Lorenzo Guerini per la preziosa collaborazione. Il sesto asse riguarda la *governance* del piano di vaccinazione, che verrà assicurata costantemente dal coordinamento tra il Ministero della salute, la struttura del Commissario straordinario, le Regioni e le Province autonome. Nella fase iniziale della campagna vaccinale si prevede una gestione centralizzata della vaccinazione, con l'identificazione di siti ospedalieri o peri-ospedalieri e l'impiego di unità mobili destinate alla vaccinazione delle persone impossibilitate a raggiungere i punti di vaccinazione. Il personale delle unità vaccinali sarà costituito da un numero flessibile di medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori socio-sanitari (OSS) e personale amministrativo di supporto. Si stima al momento un fabbisogno massimo di circa 20.000 persone. A tal riguardo si prevede di agire, da un lato ricorrendo ad un cospicuo e temporaneo ricorso alle professionalità esistenti nel Paese, anche attraverso la pubblicazione di un invito a manifestare la disponibilità a contribuire alla campagna di vaccinazione, con l'attivazione di conseguenti modalità contrattuali definite *ad hoc*, nonché alla stipula di accordi con il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei percorsi formativi delle scuole di specializzazione medica. È quest'ultima una scelta qualificante, per la quale mi corre l'obbligo di ringraziare il Ministro dell'università e della ricerca, Manfredi. *(Applausi)*. Migliaia di giovani laureati in medicina, Migliaia di giovani laureati in medicina, iscritti ai primi anni delle scuole di specializzazione, per un lasso di tempo che stiamo definendo, parteciperanno alla campagna vaccinale, che rappresenterà una parte del loro percorso formativo. Sul piano organizzativo, a livello nazionale saranno definite le procedure, gli *standard* operativi e il *layout* degli spazi per l'accettazione, la somministrazione e la sorveglianza degli eventuali effetti a breve termine. A livello territoriale verranno stabilite la localizzazione fisica dei siti, il coordinamento operativo degli addetti, nonché il controllo sull'esecuzione delle attività. A livello regionale e a livello locale saranno pertanto identificati i referenti, che risponderanno direttamente alla struttura di coordinamento nazionale e si interfacceranno con gli attori del territorio, a partire dai Dipartimenti di prevenzione, per garantire l'implementazione del piano regionale di vaccinazione e il suo accordo con il piano nazionale di vaccinazione. Con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala, *walk-in* per la popolazione, presso centri vaccinali organizzati in fase avanzata, accanto all'utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre di più la normale filiera tradizionale, incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, della sanità militare e dei medici competenti delle aziende. Il settimo asse è costituito da un moderno sistema informativo, per gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione. Per la realizzazione delle attività del piano si sta predisponendo un sistema informativo efficiente ed interfacciabile con i diversi sistemi regionali e nazionali, per poter ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali, a partire dalle forniture, fino alla programmazione e gestione delle sedute vaccinali. Inoltre, dovranno essere garantite funzionalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in particolare relativamente al sistema di chiamata attiva, prenotazione, alla registrazione e certificazione della vaccinazione, al sistema di *recall* e al calcolo puntuale in *realtime* delle coperture vaccinali e all'integrazione con i sistemi regionali e nazionali di vaccino vigilanza e sorveglianza epidemiologica. L'ottavo asse, e mi avvio alle conclusioni, un'efficace farmacosorveglianza e una sorveglianza immunologica per assicurare il massimo livello di sicurezza nel corso della campagna di vaccinazione. L'obiettivo fondamentale è quello di predisporre una sorveglianza aggiuntiva sulla sicurezza dei vaccini stessi, monitorando gli eventuali eventi avversi ai nuovi vaccini Covid nel contesto del loro utilizzo reale, identificare e caratterizzare prontamente eventuali nuovi rischi ancora non emersi ed individuare eventuali problematiche relative alla qualità. Le attività di sorveglianza saranno pianificate accuratamente in termini sia di raccolta e valutazione delle segnalazioni spontanee di sospetta reazione avversa - farmacovigilanza passiva che di azioni proattive attraverso studi e progetti di farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia. L'AIFA, in aggiunta alle attività di farmacovigilanza che sono normalmente previste per farmaci e vaccini, promuoverà l'avvio di alcuni studi indipendenti post autorizzativi sui vaccini Covid. L'AIFA si doterà inoltre di un comitato scientifico che, per tutto il periodo della campagna vaccinale, avrà la funzione di supportare l'Agenzia e i responsabili scientifici dei singoli studi nella fase di impostazione delle attività, nell'analisi complessiva dei dati che saranno raccolti e nell'individuazione di possibili interventi. Assieme alla vaccinovigilanza sarà molto importante la sorveglianza immunologica, che consentirà di valutare la risposta immunitaria indotta dal vaccino ai diversi gruppi di popolazione. Cari colleghi, spero sia risultata evidente, dalle informazioni che vi ho fornito, la portata e la complessità della campagna di vaccinazione che stiamo organizzando. Si tratta, da tutti i punti di vista, di uno sforzo senza precedenti che richiederà un grandissimo impegno collettivo. Avremo bisogno di coinvolgere puntualmente tutti i nostri concittadini per assicurare trasparenza, serietà e massima sicurezza a tutti. Non possiamo sottovalutare nessun aspetto scientifico, logistico o organizzativo. E sono certo che in un clima positivo ed unitario tutte le istituzioni repubblicane saranno in grado di svolgere un ottimo lavoro. Dobbiamo operare e lavorare tutti insieme per assicurare il pieno successo della campagna di vaccinazione per sconfiggere definitivamente questo terribile virus e per creare le condizioni sanitarie per far ripartire l'Italia. Siamo un grande Paese, non dobbiamo dimenticarlo mai. Dimostriamo ancora una volta di essere all'altezza delle sfide più difficili.

posso dire con speranza? - in generale affinché il buon senso prevalga su ogni considerazione, affinché si rimetta ordine tra le priorità e si esca dalla confusione - Natale sì, Natale no e vengano emanate quelle linee guida chiare e definitive che consentano alle persone di seguire le regole in maniera certa, senza sentirsi sempre sballottati. Ci rivolgiamo a lei affinché ci si concentri particolarmente sulla medicina del territorio (e sarebbe proprio ora), sugli operatori, sui tecnici delle ATS e delle ASST, affinché tutti - dico tutti - i professionisti della sanità vengano considerati nello stesso modo e possano collaborare, ad esempio, alla somministrazione dei vaccini nelle farmacie. Oggi lei ci ha detto che anche gli studenti di medicina la potranno fare, e noi rilanciamo chiedendo di togliere il test d'ingresso alla facoltà, sostenendo l'università. In particolare, mi soffermerò sulla questione della riapertura delle scuole al più presto, per dire no, fortemente no, al realizzarsi di una condizione contro la quale ci batteremo fino all'ultimo respiro: che non si arrivi mai a parlare di una generazione Covid. Probabilmente non ci siamo mai accorti dell'importanza della scuola come da quando si è stati costretti a chiuderle per l'emergenza; anche se dire

lo sviluppo dell'interazione con l'altro, con l'adulto, con l'insegnante, con il coetaneo, con i compagni, mentre si sono sviluppate reazioni di chiusura e vere e proprie sindromi di isolamento e di dipendenza da *computer* e cellulare. Qui però arrivano le considerazioni per il Governo, signor Ministro. Un Governo che a tutt'oggi non è stato in grado di garantire un'adeguata continuità scolastica ai nostri giovani, disperdendo la propria azione in interventi sbagliati, coprendo le falle del sistema dell'istruzione nazionale con la coperta corta della DAD, che ha aiutato a deviare l'attenzione dalle falle di un sistema che ha rivelato, e ancora non ha risolto, il problema soprattutto della mancanza di insegnanti tradizionali e di sostegno, piuttosto che affidarsi immediatamente alla scuola, subito pronta, piuttosto che avviare immediatamente un tavolo permanente di concertazione tra Ministeri della salute, dell'istruzione e dei trasporti con il Parlamento, come vera *task force*. questo al fine di evitare la riapertura e la richiusura a causa della seconda prevedibile ondata, provocata anche e soprattutto da un inadeguato sistema del trasporto pubblico, che sarebbe bastato potenziare con l'ausilio del trasporto privato, evitando dei ristori in più *(Applausi)* e usandoli

alle famiglie per scegliere la propria scuola, attuando la libertà di scelta educativa e scongiurando il pericolo delle "classi pollaio" che tanto stanno facendo discutere. siamo ancora a "caro amico virgola" e si sente parlare di far andare gli studenti a scuola la domenica. E non lo dice il ministro dell'istruzione Azzolina, ma quello dei trasporti De Micheli, che peraltro continua ad affermare che a lei nessuno ha detto che il virus si diffonde sui mezzi di trasporto. *What else*? Si sente parlare di scuola da riaprire a una settimana delle vacanze di Natale, oppure no; riapriamo il 7, ma non si sa. L'ultima notizia è che a decidere saranno i prefetti, di concerto con i sindaci. Mentre, per noi, regole, turni mattina-pomeriggio e trasporti sarebbero la soluzione. Quindi, ancora una volta, siamo di fronte a un Governo che decide di non decidere, con Ministri che demandano in continuazione a Regioni, a prefetti, a *task force*. E pensare che sono proprio i Ministri cinquestelle quelli più deleganti; proprio loro che affermano che lo Stato deve accentrare tutto su di sé. Forse

a lei oggi. Dica alle sue colleghe De Micheli e Azzolina che i ragazzi ci guardano e quello che vedono non è bello. Parlatevi e ascoltateci; ascoltateci e parlatevi. Uniamo le forze, diamo speranza al Paese perché, come dico sempre - e mi scuso per il continuo gioco di parole - la speranza è il vaccino più potente. In abbattete i pregiudizi e gli steccati; lavoriamo tutti insieme affinché la campanella di questo nuovo anno scolastico possa suonare davvero definitivamente dopo le vacanze di Natale, che auspichiamo veramente possano essere impiegate per una riorganizzazione seria e di concerto, che riporti alla normalità perché, quando la scuola tornerà a funzionare bene, sarà il segno che il Paese sarà guarito.

emergenza che è costata la vita a tanti italiani, specie a quelli più fragili, in balìa dell'improvvisazione disarmante del Governo di cui lei fa parte.

niente è stato fatto successivamente per evitare che l'onda lunga virale aggredisse le strutture ospedaliere, con la completa paralisi anche delle attività cliniche non Covid, come tutta la patologia oncologica, che pagheremo a caro prezzo. Ogni Stato avrebbe dovuto dotarsi di un piano strategico per limitare il rischio che il contagio dilagasse, imponendo con celerità interventi drastici e questo coraggio in Italia non La mancanza di protocolli e linee guida nazionali per gestire l'emergenza si è avvertita nella risposta confusa del sistema sanitario. La scelta di chi sottoporre ai tamponi ha seguito le strategie più disparate, talvolta finendo per lasciare senza diagnosi persone con sintomi evidenti e i loro familiari. I medici di base non sono stati coinvolti nella gestione della sanità territoriale e per molti giorni non si sono allestiti percorsi ospedalieri separati per i pazienti affetti da Covid, cosicché gli stessi ospedali sono diventati focolai di contagio. Il Governo ha adottato i primi provvedimenti soltanto il 23 febbraio, in presenza di 130 contagi, con l'istituzione della zona rossa del lodigiano, ma il 27 febbraio i contagi erano già 400. Eppure, mentre la curva epidemica cominciava a impennarsi, la comunicazione politica prendeva la direzione opposta, con la campagna «Milano non si ferma» promossa dal sindaco Sala e con l'aperitivo galeotto di qualche esponente politico della maggioranza. L'8 marzo i casi erano oltre 7.000 e due giorni dopo è stato dichiarato il *lockdown* nazionale, anche se secondo gli esperti, proprio quelli del suo Governo, signor Ministro, era già troppo tardi. In un'intervista al «The New York Times» Walter Ricciardi ha raccontato che lei, signor Ministro, ha faticato non poco per convincere i colleghi dell'Esecutivo ad agire più in fretta e ammette che si sono persi dieci giorni prima di fare ciò che si doveva, ma dieci giorni sono un'eternità di fronte a un virus che si diffonde così velocemente. Anche il tanto millantato apprezzamento internazionale nei confronti della gestione italiana della pandemia ha del singolare. Gli esperti della «Harvard Business School» hanno puntato il dito sulle tempistiche dei decreti adottati dal Governo per arginare il contagio, il contagio, concludendo che l'Italia ha inseguito la diffusione del virus piuttosto che prevenirla *(Applausi)*, un'analisi confermata anche dal «The New York Times» che osserva come, nei suoi tentativi di interrompere il contagio, adottati uno per volta, l'Italia si è sempre trovata un passo indietro rispetto alla traiettoria mortale del virus. In altre parole, nella gestione dell'emergenza, anziché agire in modo proattivo, si sono inseguiti gli eventi, arrivando sistematicamente in ritardo. è che, nel corso dell'emergenza, è emersa una grave difficoltà di coordinamento: la mancanza di una strategia condivisa tra diverse istituzioni coinvolte, che è sfociata in uno scontro aperto con le Regioni e qui voglio citare l'esperienza della mia Regione, la Sardegna, il rifiuto da parte del Governo della richiesta della mia Regione - che a giugno aveva debellato il virus, con un indice Rt pari a 0,03 di istituire quella che per noi era una certificazione sanitaria per garantire accessi sicuri, sia per i residenti che per i milioni di turisti che visitano d'estate la nostra terra, a garanzia di un controllo reale della circolazione virale e per mettere in protezione un sistema sanitario fragile, tarato per 1,6 milioni di abitanti. I risultati di questo rifiuto si sono visti con una recrudescenza in Sardegna del Covid-19 di importazione, salvo poi dipingere la nostra isola da parte della stampa di regime come una Regione di untori. Vedi le tre puntate di «Report» dedicate sull'argomento. *(Applausi).* E quindi, oltre al danno alla salute e all'economia, anche la beffa! Solo ora che siamo in piena fase due della pandemia il Governo cerca una condivisione con le opposizioni nel nome degli interessi degli italiani, come se noi in questi mesi fossimo stati dei semplici...

che posizione tenere e come vogliamo guardare i prossimi mesi. Di problemi, infatti, nei mesi scorsi ne abbiamo avuti abbastanza e ho già sentito un paio di interventi che sinceramente non vanno nella direzione di cui tutti abbiamo bisogno. bisogno. Sono una persona molto pacata e costruttiva, però sentire da chi governa la Regione Lombardia da vent'anni che il problema della gestione della pandemia in Lombardia sono le dichiarazioni del sindaco Sala

ma per farle funzionare e riaprirle il prima possibile hanno bisogno di un intervento di sistema dove ognuno faccia la propria parte. Bisogna anche finirla con la caricatura di cui abbiamo discusso per mesi dei banchi con le rotelle perché non è vero:

che hanno lavorato in questa direzione, però è chiaro che ancora molte cose vanno sistemate perché la scuola non finisce all'ingresso dell'aula. Ci sono ancora molti interventi da fare e c'è un tema che riguarda, in particolare, l'arrivo dei ragazzi nelle scuole. E quest'ultimo è un tema complesso perché incrocia le responsabilità nazionali con quelle regionali e comunali. Ho piacere che la collega che non vedo più in Aula

facciamo un danno perché non c'è niente di più sbagliato che fare parti uguali tra diseguali. L'unico modo di far funzionare la scuola italiana nella pandemia e - mi spiace dirlo - anche fuori è fare le differenze, valorizzare le autonomie e dare di più a chi ha più bisogno. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti perché nessuno di noi è antimodernista. Noi vediamo nella didattica a distanza anche un'opportunità, naturalmente se la si usa per fare scuola anche in maniera diversa. Questo è un tema pedagogico che non è oggetto della discussione di questa mattina, ma che ci interessa. La relazione è, però, l'aspetto più importante della scuola. La sfida incredibile

tutte le scuole in cui ciò è possibile il prima possibile; ma non possiamo sbagliare, non possiamo fare atti simbolici, non possiamo fare atti scenografici. Dobbiamo fare le cose per bene e per farlo dobbiamo fare la differenza; dobbiamo permettere di aprire a tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo, ma dobbiamo fare in modo, con rigore, che in tutti i posti in cui ciò non è possibile non si apra, non si faccia partire una catena del contagio, non si torni all'inizio della dinamica anche delle nostre scuole. Noi abbiamo una grande responsabilità, che riguarda il futuro di questo Paese e le future generazioni; questa responsabilità dipende anche, colleghi (perché ognuno

nelle case dei cittadini e che hanno la responsabilità delle proprie parole, perché il loro intervento fa opinione e che oggi vorranno sorprenderci, per la prima volta dall'inizio di questa pandemia, nell'intervento che faranno oggi in quest'Aula

il colpevole a cui dare una colpa facile per le prossime settimane, che non abbiamo in mente l'andamento dei sondaggi dei prossimi mesi o dei prossimi anni, ma che siamo impegnati a ricercare il modo in cui il Paese possa ritrovare una serietà, una responsabilità e anche una credibilità delle istituzioni agli occhi dei ragazzi. Signor Presidente, nelle scorse settimane ho parlato con tanti di questi ragazzi, che si sono trovati fuori dalla scuola a seguire le lezioni o nelle piazze, rispettando le regole. Trovo che sia straordinario che alcuni studenti, quando la scuola è chiusa,

in questo clima di chiamata generale alla responsabilità da parte di tutti e anche di collaborazione che si vuole attivare, non solo tra la maggioranza e l'opposizione, ma anche tra il Parlamento e il Governo, davanti a questa chiamata così forte a controllare in modi nuovi e anche più consapevoli la pandemia che ci ha preso e che ci tormenta da un anno a questa parte, non posso non riappellarmi direttamente a ciò che in medicina costituisce la la prima forma di cura, cioè la prevenzione. Noi sappiamo che coloro che sono morti per questa pandemia molto spesso avevano anche delle patologie pregresse, delle patologie pregresse, che riguardavano spesso il sistema cardiorespiratorio. Diciamo che questa polmonite atipica devastante, che ha prodotto tante vittime nel mondo intero, aveva buon gioco davanti a polmoni già sofferenti a causa di pregresse patologie.

L'Italia è stata il Paese che per primo, con la legge Sirchia, circa vent'anni fa, si è dotato di uno strumento di prevenzione delle patologie, sia di tipo infettivo, sia di quelle connesse a una sorta di degenerazione del tessuto polmonare, sia di tipo oncologico. noi abbiamo assistito, da pochissimi anni a questa parte, a un'operazione menzogna, che ha cercato di sostituire il fumo classico (chiamiamolo così) con il cosiddetto tabacco riscaldato. È un'operazione menzogna, devo dirlo al Ministro, quale fa verità la lettera recentemente pubblicata dal suo direttore generale alla prevenzione, il dottor Rezza, a tutti gli assessori regionali. Fa verità perché afferma cose importanti: che

convincendoli che, cambiando modello di sigaretta, avrebbero potuto recuperare addirittura qualità di vita - la peggiore delle risposte che il Governo potesse dare è stata quella che tutti conosciamo: lo sconto fiscale. Attenzione, in questo momento la notizia fa scandalo e lo dico agli amici del MoVimento 5 Stelle, perché fa scandalo la commistione che ci potrebbe essere,

scandalo (lasciamo che se ne faccia carico la magistratura), ma del danno certo alla salute e dell'aggravamento forte che questo comporta per i fumatori cronici che decidono di smettere di fumare e per i giovani adolescenti che cominciano a farlo. Per questo facciamo appello al Ministro della salute, perché non si può agire soltanto sulla distanza fisica, sulla mascherina e sul *gel* - tutte cose sante e benedette - ma bisogna farlo più a monte, mantenendo la salute dei nostri polmoni nelle migliori condizioni possibili, e il fumo è devastante. è devastante. Dobbiamo avere il coraggio, allora, di dire qualcosa di più quando parliamo di prevenzione. Sicuramente possiamo far riferimento all'inquinamento atmosferico, che pure è uno dei fattori che comportano disagio e sofferenza a tutte le nostre funzioni respiratorie, ma il fumo è una delle cause più conclamate e più chiare,

ristori che possono addolcire la fatica, e non devono subire questo danno - che a noi sembra un vantaggio per la salute di tutti gli italiani - ad esempio le aziende produttrici di tabacco?

e chiusuristi, che sta raggiungendo forse il massimo livello del surreale. Assistiamo ancora, dopo tutto quello che è successo, a dibattiti interminabili e senza soluzione tra virologi che, in realtà, fino a qualche tempo fa erano ignoti anche ai loro pazienti. Vediamo discussioni da salotto ovunque e abbiamo assistito anche alla penosa storia della scelta del commissario alla sanità in Calabria, che, se non fosse un'autentica tragedia, in un film potrebbe anche far sorridere. Dobbiamo prendere atto che il dibattito pubblico forse non è all'altezza della sfida che il nostro Paese è chiamato a sostenere e che il dibattito parlamentare è stato completamente esautorato sul tema e confinato.

quasi 500.000 piccole imprese a rischio chiusura. E siamo qui a varare un decreto-legge alla settimana rincorrendo le istanze, i vuoti e le dimenticanze, nell'ottica della teoria della rincorsa, piuttosto che della strategia. Ricordate che il futuro dovrà sopportare il peso di un debito pubblico che mai abbiamo avuto, dal Dopoguerra in poi. Il futuro vedrà l'Italia confidare nella capacità delle imprese di lavorare, creare posti di lavoro e reggere la crisi economica. Il Governo deve capacitarsi di tutto ciò. Queste sono scelte da farsi quando si ha un piano, ma la questione è che esso è mancato. L'Italia poteva forse evitare l'impatto della seconda tornata. Avevamo anche i dati disponibili, ma tutto è stato consumato in una drammatica esperienza, dalle mascherine alla riapertura delle scuole, con i famosi banchi a rotelle, i trasporti, il sistema dei test, il tracciamento e il trattamento.

era facile prevedere che, con la riapertura delle attività scolastiche, si sarebbero potute determinare inevitabili criticità. Il Presidente della Regione Lombardia ha scritto al ministro Boccia, anticipandogli che il regolare avvio dell'anno scolastico, secondo calendario e modalità consuete, avrebbe reso insostenibile la conseguente domanda di trasporto.

ringraziare il ministro Speranza per le comunicazioni in riferimento al DPCM che elenca le misure che diventeranno effettive da questa settimana fino alla fine del periodo natalizio. È importante sottolineare la grande responsabilità con la quale il Governo sta affrontando la crisi pandemica e il grande realismo con il quale prende le importanti decisioni contenute nei provvedimenti emanati. È ovvio che, come italiani, non possiamo che essere, da un lato, preoccupati e, dall'altro, infastiditi per alcune limitazioni alla nostra libertà di spostamento sul territorio nazionale. però certo che, come cittadini, sentiamo anche sulle nostre spalle tutto il peso della responsabilità di uscire al più presto dalla pandemia. Dobbiamo essere ben consci che la nostra libertà personale finisce dove inizia il diritto del prossimo alla salute e, in alcuni casi, anche alla vita. Questo perché, se a molti il virus non ha comportato alcun tipo di danno, a tanti nostri concittadini, magari anche parenti, può aver portato gravi complicazioni, senza dimenticare che la pandemia ha portato alla morte oltre 50.000 persone. Succede vediamo i classici detrattori, i complottisti, gli sciamani e gli stregoni da piazza, quelli del "la verità la so io", i bufalari da *social network*, fare più danni dello stesso virus. stesso virus. Dobbiamo ritrovare un profondo spirito di unità nazionale, quello che il nostro Paese ha saputo risvegliare, ad esempio, dopo le più brutte pagine della nostra storia, come le grandi guerre mondiali. In quei precisi periodi storici l'Italia veniva fuori dalle macerie e forse la differenza è proprio questa: a quel tempo, gli italiani, almeno la maggior parte di loro, avevano poco o nulla e quel poco però era sufficiente per stringersi intorno a uno spirito nazionale, che rendeva orgogliosi di sentirsi italiani; oggi il mondo è cambiato, l'economia ormai è globalizzata e sicuramente il nostro tenore di vita è completamente diverso da allora. Per questo per molti è così difficile anteporre la salute agli interessi meramente economici, personali. allora che l'onere delle decisioni ricada sul Governo e sul Parlamento. Fino a oggi non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle nostre responsabilità, a partire dalla responsabile scelta di contemperare gli interessi economici con quello primario della salute. Chi è dotato di onestà intellettuale non può che riconoscere all'Esecutivo la ferrea volontà di non chiudere nulla che non fosse strettamente necessario. Certo, l'eccesso di zelo a volte non paga e voglio esprimere qui l'auspicio che le scuole riaprano tutte al più presto: solo perché non sono un'attività economica, non vuol dire che non siano altrettanto importanti; tra l'altro le superiori sono al momento chiuse, non tanto per un problema di contagi al loro interno, del tutto risibile, ma a causa dell'organizzazione del trasporto pubblico. non possiamo permetterci di continuare a lasciare i ragazzi a casa: un intero anno scolastico senza didattica in presenza avrebbe conseguenze drammatiche, specialmente sulle classi sociali più esposte in questa crisi. Proviamo a riaprirle in sicurezza già questo mese: questo sì che sarebbe un ottimo segnale, anche parziale; proviamoci! Tante attività economiche sono state coinvolte dalla pandemia. Si è cercato di limitare solo quelle in cui il contatto interpersonale è inevitabile veicolo per il *virus.* Nonostante questo approccio, molto pragmatico, ogni giorno leggiamo sui giornali una lotta tutta politica di questo o di quel partito che prende le parti di un settore economico. Vorrei ricordare che, da quando è scoppiata la pandemia, Governo e Parlamento hanno contribuito ad approvare ben nove provvedimenti; abbiamo stanziato 100 miliardi di euro di *deficit*, gran parte dei quali destinati alla tutela dei lavoratori e ai contributi a fondo perduto per le attività economiche. Con gli ultimi quattro provvedimenti (ovvero il pacchetto dei decreti-legge ristori), abbiamo messo in campo 18 miliardi di euro per aiutare le attività più colpite, in conseguenza della divisione del Paese in zone di rischio, e per dare respiro al nostro tessuto economico-produttivo, con una vasta serie di proroghe fiscali. È *in itinere* una manovra da 40 miliardi, che ne stanzia quattro per futuri indennizzi a fondo perduto, ai quali si aggiungeranno presto le risorse di un quinto decreto-legge ristori, che andrà incontro alle imprese che hanno subito cali di fatturato, pur non avendo direttamente chiuso. In tutto questo, naturalmente, massima attenzione è stata data alla sanità. Dall'inizio di questa emergenza, abbiamo stanziato quasi 10 miliardi; abbiamo potenziato il Servizio sanitario nazionale, prevedendo aumenti di posti letto, assunzione di medici e infermieri, indennità aggiuntive, potenziamento della medicina territoriale e tanto altro ancora, ma scontrandoci purtroppo con i limiti della riforma del Titolo V della Costituzione, per cui all'azione del Governo non tutte le Regioni hanno risposto in modo adeguato. Se ne parlava proprio la scorsa settimana, durante la discussione sullo scostamento di bilancio. Non c'è chi non veda in tutto questo la quantità e la qualità dello sforzo profuso. Colleghi, per cortesia, evitiamo toni e modi da campagna elettorale: l'Italia Siamo in inverno, una stagione in cui, come tutti sappiamo, intere aree alpine e appenniniche attendono la neve, perché vivono di sci e, in generale, di turismo legato agli sport invernali;

È troppo alto il rischio di buttare tutto all'aria. Se lo sci è uno sport individuale che si fa all'aria aperta, tutto ciò che gli ruota intorno, dalle soste in baita alle code per noleggiare attrezzature, dagli *skipass* all'accesso agli impianti, può creare pericoli. È chiaro che un'eventuale chiusura non ci lascia indifferenti: interi Comuni montani vivono esclusivamente di questo; la montagna è PIL, lo sappiamo benissimo, per questo, come MoVimento 5 Stelle, ci prenderemo in carico l'onere di una decisione così sofferta, individuando il meccanismo migliore per risarcire tutti gli operatori di questa filiera interessati da un eventuale stop. Lo abbiamo fatto per tanti segmenti del nostro mondo produttivo e lo faremo anche stavolta, senza tentennamenti e col massimo sforzo. Non è possibile però replicare l'errore dell'estate, quando si è voluto ascoltare i gestori di locali e discoteche per dar loro una *chance.* Tutti abbiamo visto come hanno gestito questa possibilità: locali stracolmi, mascherine abbassate o del tutto assenti, contagi che hanno proliferato tra clienti e personale dei locali. Un noto imprenditore della Costa Smeralda, rispondendo alla stampa sulle proprie mancanze, si è giustificato dicendo qualcosa del tipo: mica potevamo sparare alla gente. Sparare no, non sarebbe servito; bastava farne entrare meno e controllare il rispetto dei protocolli Per questo passeremo un Natale solo con gli affetti più cari, ma che siano pochi. Non potremmo perdonarci la colpa di contagiare qualcuno più debole di noi. Chi ha il dono della salute ha anche la responsabilità di preservare quella degli altri

il ministro Speranza ha ricordato in quest'Aula che sono molti i candidati vaccini, attualmente in studio: sono 157, di cui 88 in fase preclinica, 40 in fase clinica 1, 17 in fase clinica 2, 13 in fase clinica 3, la più avanzata. Ebbene non uno di questi, non uno, avrebbe potuto procedere o procederà senza sperimentazione animale. Il che significa che, senza sperimentazione animale, non avremo mai un vaccino o una cura che ci permetta di sconfiggere Sars-Cov-2. Poiché l'ignoranza dei fatti è un alibi pericoloso, che condanna chi se ne alimenta ad una percezione distorta della realtà, vorrei qui ripercorrere brevemente, a titolo di esempio, l'apporto della sperimentazione animale negli studi per ottenere il vaccino dell'americana Moderna,

e quello che studia nei topi lo fa grazie ai vent'anni pregressi di ricerca su topi, furetti e conigli. Arriva a ottobre, quindi due mesi fa, la sua pubblicazione sul «New England Journal of Medicine», dal titolo autoesplicativo «Valutazione del vaccino mRNA-1273 in primati non umani», quindi nei macachi. Sono dodici i macachi impiegati per ogni sesso, tra i tre e i sei anni. Sono selvatici, hanno maggiore similarità all'uomo per gli aspetti di replicazione del virus nelle vie aeree e dell'immunologia, mediata da cellule T e B, che i roditori non hanno. Gli scienziati di Moderna sottolineano che l'impiego dei macachi permette di studiare la scalabilità del vaccino, quindi quali dosi di vaccino siano

a proposito dell'apporto della sperimentazione animale, che cos'è successo e quali sono stati i passi per conoscere e affrontare questo virus, con un vaccino che lei, signor Ministro, riprendendo la definizione della Commissione europea, ha chiamato "bene comune". Concludo davvero chiedendo a tutti, in quest'Aula, un atto di onestà intellettuale. Bisogna dire che chi si oppone alla sperimentazione animale cento della quale è condotta su topi e ratti) dev'essere consapevole che la sua posizione, se avallata dalle istituzioni, condannerebbe il mondo a soccombere di fronte a un virus, rinunciando a poterlo combattere e sconfiggere con vaccini e cure che arriveranno grazie alla sperimentazione animale condotta dai nostri studiosi, giovani e meno giovani. Mi rivolgo quindi a lei, signor Ministro, perché fin dalle prossime settimane, in un soprassalto di legittimo orgoglio per la funzione ricoperta, in un momento storico così difficile per la salute di tutti noi, sappia far prevalere sulle logiche identitarie e di riconoscibilità di partito l'interesse dei cittadini a una libera ricerca biomedica, di cui lei è chiamato per funzione istituzionale ad essere il primo responsabile.

l'approccio che ha dato oggi alle sue comunicazioni al Senato della Repubblica: evitare che la campagna di vaccinazioni possa coincidere con una nuova ondata dell'epidemia. Seguirò il suo filo: lei, signor Ministro, in nome di queste affermazioni, deve procedere a un'interlocuzione serrata con le Regioni per predisporre un piano nazionale di sorveglianza attiva, unico,

Non possiamo ignorare le sofferenze e le preoccupazioni di tanti, troppi concittadini, ancora oggi bloccati a casa a causa della mancanza dell'esecuzione di un tampone in tempi rapidi per accertare la malattia, che, se effettuato per tempo, dopo la fine della malattia, consentirebbe loro di tornare al lavoro e alla vita sociale. Quanti familiari di persone positive conosciamo, a cui non si fa un tampone e che vivono tra le mura domestiche con l'incubo del contagio? Un sistema Un sistema di tracciamento efficace è fondamentale per proteggere persone e famiglie, strutture per persone con disabilità e più fragili. Domani celebriamo la giornata della disabilità e le persone con disabilità hanno subito molto di più le conseguenze dell'epidemia. Questo piano dev'essere accompagnato da una campagna - l'abbiamo detto in Aula qualche mese fa - per rendere edotti i cittadini sui vari test e sul loro uso. uso. Signor Ministro, il fatto che a un certo punto a fine settembre si sia perso di vista il tracciamento grida vendetta, perché abbiamo lasciato le persone sole di fronte all'infezione o in fila ai *drive*-*in*. Non dobbiamo dimenticarlo. È dovere del Governo e delle Regioni - proprio adesso che la curva dei contagi sta flettendo - avere nel nostro Paese una politica di tracciamento degna di questo nome, facendo tesoro delle esperienze che hanno funzionato nella prima fase dell'epidemia e di quelle dei Paesi in cui si è contenuta nella seconda fase, ed evitare che la terza ondata ci scappi di mano; inserire il rafforzamento della sorveglianza sanitaria dentro il piano pandemico e, coerentemente con quello, per oggi e per il futuro. Dico questo proprio oggi, perché parliamo di vaccini e, come ha detto, anche della verità che abbiamo davanti a noi. La verità è che, come sappiamo tutti, almeno nei primi mesi dell'anno, non saremo in tanti a essere vaccinati e dovremo continuare a raccomandare prudenza ai cittadini, rispetto delle regole come stiamo facendo anche in occasione del Natale - ma, nello stesso tempo, rassicurare la popolazione sulla nostra capacità di sorveglianza sanitaria. Le altre cose che dovremo organizzare da subito sono l'assistenza domiciliare e la medicina territoriale, grandi assenti nella prima fase dell'epidemia, dimostrando che, laddove sta funzionando, l'accudimento domiciliare porta grandi benefici e non conduce all'affollamento degli ospedali: dobbiamo averlo averlo sempre a cuore, come diceva lei. La Commissione sanità che mi onoro di presiedere intende dare un grande contributo di idee e proposte a tale proposito, e nei due anni di legislatura che abbiamo davanti è necessario trasformare il sistema sanitario, partendo dal territorio e indicando un modello nazionale. mettere in atto, signor Ministro, non da solo, ma insieme al Governo - anche di questo abbiamo parlato tante volte in queste Aule - è un piano di trasporto locale, anche con accordi con il privato, e ogni iniziativa utile per evitare sovraffollamenti sui mezzi pubblici e assembramenti. Arriviamo ai vaccini. È molto importante quello che ci ha detto in quest'Aula. Penso che avremo un prima e un dopo Covid: individualità *versus* socialità; quindi, non bisogna vedere la società come compartimenti stagni (gli anziani, i fragili e tutti gli altri), perché siamo un insieme. Dovremo accompagnare la popolazione, informandola sull'importanza dei vaccini, proprio per proteggere i più deboli e rendere consapevole la cittadinanza che questo virus è meglio non prenderlo. Sarà necessario arrivare al 70 per cento di immunità di gregge per tornare alla vita normale; di questo tutti abbiamo un gran desiderio. medicines agency (EMA) stanno conducendo una partita importantissima sui vaccini, come ricordava lei. Ieri abbiamo tenuto un'audizione con la dottoressa Gallina, che ci ha rappresentato anche i valori di fondo che l'Unione europea

penso si debba anche valutare un nuovo studio sierologico, per capire anche la vera prevalenza del contagio nelle Regioni e regolarsi sulle vaccinazioni. Questa nuova fase, signor Ministro, dovrà essere all'insegna della consapevolezza, della preparazione, dell'informazione, della trasparenza e delle non contraddizioni.

Signor Presidente, ringrazio il ministro Speranza per il suo esaustivo intervento, in cui ha spiegato lo stato dell'arte. È vero che i vaccini anti-Covid rappresentano finalmente una speranza concreta per uscire dal *tunnel* della pandemia. Dalla comparsa del Covid-19, alla fine dello scorso anno, la ricerca medica, sia pubblica sia privata, si è attivata come mai nella storia, producendo risultati di conoscenza, messa a punto di protocolli terapeutici e anche diversi candidati vaccini, che sembrano garantire una protezione, a seconda dei comunicati delle aziende, per oltre il 90 per cento dei vaccinati, apparentemente con assenza Come ci ha spiegato il signor Ministro, la corsa al vaccino è stata possibile in tempi così brevi non solo per la grande entità degli investimenti, ma anche per l'attivazione, da parte delle agenzie di controllo, di una modalità speciale, chiamata *emergency use authorization*, ovvero un'autorizzazione per uso emergenziale, che, come ci ha spiegato il Ministro, ha visto le varie fasi cliniche concentrate in parallelo, anziché in serie. Quest'autorizzazione viene rilasciata in situazioni emergenziali, sulla base di un calcolo tra rischio e beneficio che ne giustifichi il rilascio. Non serve argomentare quanto sia opportuno attivare una procedura autorizzativa di questo tipo, quando il virus ha causato già più di 50.000 decessi solo in Italia e quasi un milione e mezzo nel mondo. La durata minima della sperimentazione in fase 3 del vaccino, per determinare sicurezza ed efficacia in modalità emergenziale, tuttavia, è di soli due mesi dalla seconda immunizzazione. Non bisogna dimenticare, come ha ricordato il Ministro, che questo tipo di autorizzazione, peraltro non ancora rilasciata per nessuno dei candidati vaccini anti-Covid,

Probabilmente ci vorranno mesi prima che qualsiasi vaccino per il Covid-19 ottenga la piena approvazione delle agenzie regolatorie, condizione ineludibile per una campagna massiccia. in questo periodo, come ha ricordato il Ministro, non si può abbassare la guardia ed è ancora necessario avere misure di contenimento, di limitazione degli spostamenti e di attenzione,

Ben venga perciò il piano di distribuzione dei vaccini che il Ministro ci ha illustrato, che dev'essere accompagnato, come giustamente ha dichiarato, da una corretta informazione, ma anche da un attento e complesso monitoraggio dei vari candidati vaccini, perché ad oggi non sappiamo ancora quale sarà il più efficace e il più sicuro. Ci sono domande a cui la comunità scientifica non ha ancora dato risposte, che solo da questa prima fase di vaccinazione impareremo e che non ci consentono di abbassare la guardia, *in primis* sulla durata della protezione. Come ha detto il Ministro, non è nota e non sappiamo se i vaccinati la manterranno a lungo. Non meno importante - su questo vorrei insistere, perché la comunità scientifica ne ha molto discusso - è il tema della possibile contagiosità dei vaccinati, nel caso contraggono il virus dopo la vaccinazione.

È molto probabile che ci troveremo in una situazione intermedia, ove alcuni vaccinati saranno non infettivi, mentre potrebbe succedere che altri, se si infettano, diventino a loro volta infettivi. Su questo non possiamo trarre conclusioni finché non avremo fatto le dovute verifiche nei prossimi mesi.

Prescindendo dalla discussione sulla trasparenza dei dati che anima il mondo scientifico in queste settimane, che tuttavia non compete a quest'Assemblea legislativa, perché i dati scientifici li deve analizzare chi è capace di farlo, farlo, non dobbiamo dimenticare che il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini non può basarsi sugli annunci delle case produttrici, ma deve prevedere trasparenza, tutela e controllo continuo da parte del Governo. L'esitazione vaccinale è un fenomeno complesso e difficile da affrontare e non si può liquidare con un "vaccinatevi tutti, altrimenti siete degli sconsiderati". È uno dei pericoli globali per la salute pubblica del 2019, secondo l'OMS. Un italiano su sei ha già deciso che non si vaccinerà,

impensabile per un vaccino autorizzato in fase emergenziale, di cui ancora si deve valutare la sicurezza. Non si può obbligare un cittadino a vaccinarsi in questa fase, ma anche dopo la fiducia si dovrà conquistare, non si potrà imporre, quindi sarà altrettanto importante costruire, in questi mesi che precedono l'autorizzazione definitiva, un percorso inclusivo e trasparente, affinché l'obbligo diventi morale per i cittadini e ci sia la fila per vaccinarsi. Per questo spero che la risoluzione di maggioranza abbia incluso raccomandazioni in tal senso. Se da un lato, però, stiamo per affrontare un percorso di monitoraggio e persuasione al vaccino,

La pandemia, come ha dichiarato l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), rappresenta una devastazione senza precedenti non solo per la salute, ma anche per l'economia globale e il commercio. L'emergenza sanitaria prodotta dal nuovo coronavirus richiede, come mai prima, condizioni di accesso rapido a tutti gli strumenti medicali, inclusi prodotti farmaceutici come diagnostici, vaccini e farmaci per la prevenzione del contagio e la cura delle persone malate. La scarsità colpisce soprattutto (ma non solo) i Paesi a medio e a basso reddito, mette in grave pericolo di vita il personale sanitario di tutto il mondo - non solo del nostro Paese - e determina il decesso di un numero significativo di lavoratori essenziali durante questa prolungata pandemia. Sin dall'inizio della pandemia, la possibilità di accesso ai prodotti essenziali nel mondo è fortemente disuguale, non è uguale per tutti. Alcuni rifiutano il vaccino e altri purtroppo non lo possono avere. I Paesi più ricchi, che rappresentano il 13 della popolazione mondiale, si sono già accaparrati più di due miliardi dosi dei potenziali vaccini contro il Covid-19. Una delle principali barriere di accesso ai farmaci essenziali risiede nei diritti di proprietà intellettuale, ovvero nel regime di monopolio brevettuale intellectual property rights (TRIPs) dell'Organizzazione mondiale del commercio conferiscono alle industrie. Per questo il 14 novembre 2001 gli stati membri dell'OMC adottarono la storica dichiarazione di Doha che riconosceva loro la prerogativa di usare tutte le flessibilità necessarie per rispondere alle necessità di salute pubblica in deroga ai brevetti. India e Sudafrica hanno proposto di sospendere i trattati Trips ed hanno chiesto il supporto a molti Governi. Chiediamo dunque che l'Italia si adoperi con convinzione, in seno all'Unione europea, di concerto con altri Paesi, affinché l'ostilità della Commissione all'iniziativa di India e Sudafrica sia immediatamente rivista e sia invece accolta per Covid-19 la temporanea eccezione al regime ordinario dell'accordo Trips, in modo che il vaccino diventi veramente un bene comune. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere qui oggi ad informarci sulla situazione relativa al Covid, ma anche sul piano strategico di acquisizione del vaccino e sul piano di vaccinazione della popolazione. Le misure adottate nei precedenti DPCM hanno portato ad intravedere risultati positivi, come lei,

ai conteggi che abbiamo tutti i giorni, credo che ce lo facciano tenere ben presente. Le nuove disposizioni quindi vanno in questa direzione: evitare la terza ondata - perché quello potrebbe essere il futuro che davvero non possiamo più permetterci sia dal punto di vista sanitario (la pressione sulle nostre strutture e sugli operatori sanitari, che ringraziamo sempre, non possono più andare oltre)

classificazione delle Regioni in base alle emergenze sanitaria ed epidemiologica, che cambiano in maniera estemporanea. Si tratta di un'aggiunta rispetto a quello che doveva essere un *lockdown* nazionale, e che invece ci sta aiutando a preservare alcune Regioni.

so che è stato fatto tanto, però le chiedo di insistere ancora su questo tema, perché le persone devono ricevere ascolto soprattutto nel momento in cui sono isolate ed hanno bisogno di un conforto e di parlare con qualcuno che dia loro attenzione.

che sarà il preludio per avere eventualmente una sanità unificata anche in Europa. È importante, secondo me, vedere delle opportunità che si possono cogliere in un'emergenza di questo genere.

Quindi vaccinarsi diventerà un atto di responsabilità civile per raggiungere quell'immunità di gregge di cui lei, Ministro, parlava prima. È bene che il vaccino sia un bene comune e gratuito per tutti, anche per coloro che non se lo possono permettere. Dobbiamo quindi giustamente mettere attenzione su questo.

Un'altra cosa che lei ha detto, signor Ministro, sulla quale sono molto d'accordo, è di impiegare subito i nostri laureati e i nostri futuri specializzandi per aiutarci a fare le vaccinazioni. Va benissimo,

Ci sono state delle emergenze e su queste si è intervenuti. La didattica a distanza non è la soluzione e non lo sarà mai, perché i rapporti interpersonali che si creano nelle scuole sono fondamentali e importanti per la crescita dell'individuo. Quindi, da questo punto di vista bisogna assolutamente fare di più sul tema del trasporto, che ancora non è stato risolto. Infine, signor Ministro, ci tengo a dire un'ultima cosa. I fondi purtroppo finiranno. Giustamente li abbiamo usati per contrastare e tamponare la situazione di emergenza, ma dobbiamo pensare al futuro, a rendere strutturali le assunzioni che abbiamo fatto nel nostro sistema sanitario, usando il Fondo sanitario nazionale per parte corrente, perché sappiamo che le persone vengono pagate con la parte corrente. Usiamo invece altri fondi per gli investimenti; ce ne saranno altri e devono essere usati per investire sulle case di comunità, sugli ospedali e sulla digitalizzazione. Grazie, signor Ministro: questo è il nostro pensiero.

Il Governo è arrivato fortemente impreparato alla seconda ondata, senza una strategia: è mancata una programmazione seria ed efficace; non c'è stata la giusta prevenzione. Avete avuto mesi per potenziare il trasporto pubblico, per assumere medici e infermieri, per aumentare le terapie intensive, ma nulla è stato fatto in tutto questo periodo. Si è perso solo tempo. Per diversi giorni in televisione abbiamo visto scorrere un annuncio, che iniziava con una domanda: «Sei un medico?» e terminava con un'offerta di alloggio, di un'indennità giornaliera e di un rimborso spese. Non è questo forse l'ennesimo simbolo della mancanza di quella programmazione che un Governo responsabile avrebbe dovuto porre in essere per tempo? Non avete potenziato i trasporti, così come avete potenziato il tracciamento e la medicina di base; non avete rafforzato il Servizio sanitario nazionale, eppure lo avevano detto tutti che ci sarebbe stata una seconda ondata; «Tracciamento» e «prevenzione»: queste dovevano essere le parole d'ordine. Tutti i programmi che hanno avuto successo nel contrasto al virus si sono basati sul tracciamento degli asintomatici. Siamo nell'attuale situazione perché da maggio a settembre nessuno ha messo in piedi un piano. Solo l'encomiabile lavoro di tutti coloro che hanno operato e operano sul campo, in trincea (e lo ha ricordato anche lei, signor Ministro), dagli operatori sanitari a tutti coloro che con enorme sacrificio combattono ogni giorno per aiutarci, ha permesso di evitare uno scenario ancora peggiore. L'impressione è che chi ci governa navighi un po' a vista, con un colpo al cerchio e uno alla botte: prima vieta una cosa, poi cede e la concede un po', senza un programma, senza una linea, senza nulla che ci faccia capire che cosa sia davvero meglio per il bene del Paese. La seconda ondata è purtroppo il frutto prevedibile e previsto delle omissioni dei mesi scorsi su tutti i versanti cruciali: nessuna programmazione dei tamponi dei *drive-in*, nessun tracciamento dei contatti, nessun controllo degli assembramenti, nessuna assunzione di personale sanitario, nessun rafforzamento delle terapie intensive. Anziché fare queste cose, ci avete raccontato che tutto il mondo ammirava il modello italiano di contrasto all'epidemia e ci avete dato - mi consenta la polemica banale - banchi a rotelle e monopattini cinesi.

perché il tutto solleva interrogativi gravissimi che si aggiungono ad altri mai chiariti in passato. Pretendiamo per l'interesse degli italiani parole di verità. C'è chi ha avvertito del pericolo a maggio, chi a giugno e chi a luglio, ma a partire dalla metà di agosto non si poteva non capire perché tutti gli indicatori - lo sottolineo - dicevano che la curva non cresceva più linearmente, ma esponenzialmente. Ora i nodi sono venuti al pettine e grande è la confusione. Ci sono punti di vista e posizioni diverse annunci roboanti che sono rimasti solo annunci. Proprio le singole misure governative ci mostrano quanto tardiva e quindi inefficace sia stata questa strategia. Ora vi siete ricordati di interessare i medici di base per i test rapidi e per la copertura assistenziale del territorio; ora il Governo tira fuori il suo piano per combattere il virus. Signor Ministro, nel ristori-*ter* avete messo 100 milioni di euro da dare ad Arcuri per l'acquisto di farmaci anti-Covid, ma quali sono questi farmaci visto che ieri nelle linee guida non sono indicati farmaci particolari? *(Applausi).* È tardi e, purtroppo, lo hanno capito sulla propria pelle tutti gli italiani. Signor Ministro, da mesi vi sentiamo dire che il Sistema sanitario nazionale va rafforzato, Signor Ministro, da mesi vi sentiamo dire che il Sistema sanitario nazionale va rafforzato, allora si cominci a fare qualcosa di concreto.

a carico del Servizio sanitario regionale, completata nel 2018, che sta causando e che causerà a breve il ridimensionamento di molti reparti e molte strutture ospedaliere in molte Regioni, compresa la mia e la sua. Oggi, di fronte Oggi, di fronte a una crisi sanitaria che ha duramente colpito le nostre strutture sanitarie è assurdo chiudere o ridimensionare molte di queste strutture. Signor Ministro, dite che dovremo convivere a lungo con questo virus e ciò a prescindere dai vaccini. Cosa pensate di fare? Chiuderci a casa tutte le volte perché per voi è la scelta più facile? Se questa irresponsabilità poteva anche essere giustificata a marzo, quando nessuno sapeva con cosa si aveva a che fare, quanto accaduto da settembre non ha alcuna giustificazione e nessun *mea culpa* è stato proposto dal presidente del Consiglio Conte: non ha mai chiesto scusa agli italiani. L'incapacità di organizzare e di prepararsi a una nuova ondata Covid sono l'emblema e la responsabilità di questo Governo. Ci auguriamo che ciò non accada anche per ciò che riguarda il piano vaccini, che lei ci ha illustrato,

per il comitato tecnico-scientifico i ristoranti potevano tenere aperto la sera e se, quindi, è stata una decisione presa di sua spontanea volontà senza ascoltare i tecnici con cui collabora il Ministero. notizia fosse vera, sarebbe molto grave. Prima di entrare nell'argomento, volevo ricordare che alcuni colleghi in Aula hanno parlato di necessità di collaborazione visto che siamo in

quindi a rivedere un po' le tradizioni celtiche: preferisco oggi essere considerato il Grinch piuttosto che Babbo Natale nei vostri confronti. Per fare questo intervento, signor Presidente, sono andato a riprendere un'*email* che mi è stata inviata stanotte da un imprenditore della mia città e mi piacerebbe condividerla con voi, leggendola, perché è quello che la gente, che gli italiani pensano di voi: «Caro Gianma, scusa il disturbo, ma ormai la notte dormo sempre meno e mi permetto di scriverti, come si dice, di pancia questo messaggio, come cittadino e come imprenditore italiano. Per l'Italia ti dirò una cosa scontata: maggio, giugno, luglio, agosto, quattro mesi di tregua per organizzare le cose e invece niente. In estate controlli, organizzazione e monitoraggio zero. Hanno dato regole che non hanno fatto rispettare per nulla (vedi con noi ristoratori). In autunno è arrivata la seconda ondata; prevedibile? Certo. E quindi piano scuola: fatto qualcosa? Nulla. Piano trasporti, fatto qualcosa? Nulla. Piano ospedali, fatto qualcosa? Nulla. E allora che cosa fa il Governo? Chiude. La cosa più facile: nel dubbio, chiudo tutto e non sbaglio. E quindi, dopo, la "via del Risiko", delle zone rosse, arancio, gialle, per fingere un tentativo di non *lockdown* totale, anche se nelle zone rosse le regole di base sarebbero state quelle del *lockdown* di marzo. Vuoi un esempio? Io ho fatto in macchina Milano-Roma, ho girato Roma parecchio e sono tornato: non ho mai visto un controllo. Un Governo che fa e non controlla. Fondamentalmente, nel non avere la forza di fermare tutto, veramente tutto, accorgendosi dell'imperizia estiva, si sono messi a chiudere un po' di cose e a giocare coi pastelli. intanto facciamo 700 morti al giorno. Qualcuno dirà: ma anche gli altri Stati hanno problemi. Bella soddisfazione! Ma cosa hanno fatto gli altri Stati per sostenere le aziende chiuse? Soldi, tanti e subito. Un esempio, la Germania: le misure economiche tedesche, oltre 353 miliardi di euro, più oltre 800 miliardi di garanzia sui prestiti, varati nei vari mesi, da marzo-giugno in poi. In Italia, niente. In Germania, soldi arrivati tutti e subito. Se sei al Governo, caro Ministro, devi dare delle regole, devi farle rispettare e dimostrare che le tue scelte salvano vite ed economia. E poi c'è la credibilità. Mi esci in tv e dici che fai, che dai e che fai, ma non è assolutamente vero. L'ultima su tutti: i ristori arriveranno sicuramente entro il 15 novembre. Non è vero, a me non è arrivato nulla. Non devi dire le bugie. La cassa integrazione non la devi dare dopo tre mesi, se va bene, ma la devi dare subito. I tempi e le decisioni sono fondamentali. E adesso, caro Stato, non ti credo più. Hai le scuole superiori e le università chiuse? Sì. Hai gli ospedali pieni? Sì. Avevi detto agli imprenditori di adeguarsi alle regole Covid, che poi avresti riconosciuto il 60 per cento in credito di imposta? Hai sbagliato i conti e l'hai fatto diventare circa il 16 Ma di cosa stiamo parlando? Neanche mio figlio, che ha sei anni, sbaglia così tanto un compito di matematica. Hai attività aperte in difficoltà e altre completamente chiuse. E poi decidi di tenere gli impianti sciistici chiusi, facendo un altro danno al turismo enorme perché non ti sei organizzato per tempo con regole per i comprensori? Sì. Però voglio vedere chi va in Austria o in Svizzera a sciare come li fermi e garantisci la quarantena». Questo imprenditore aggiunge: «Ho decine di amici che hanno già prenotato. Stai facendo fallire il mondo del turismo e il turismo aereo e stanno arrivando gli zampini degli speculatori internazionali sui nostri hotel. Lo sai, Governo, che stanno fallendo centinaia di ristoranti che si sono adeguati e tu non hai controllato? E adesso li tieni tutti chiusi, con migliaia di persone in cassa integrazione. Ma lo sai, Governo, che intanto nelle case e nelle taverne private si continuano ad organizzare cene e feste senza nessuna regola? E, fidati, se vuoi ho un elenco di cinque pagine scritte in piccolo. Il Governo ha saputo evitare tutto questo? No. Muoiono 700 persone al giorno? Sì. E allora il Governo ha fallito. Punto». La lettera di questo imprenditore io la sottoscrivo in pieno, perché fa una fotografia di quello che sta succedendo ed è successo in questo Paese. *(Applausi)*. Non state governando la pandemia; non state governando nulla! E adesso, Ministro, ci dite che a Natale gli italiani non potranno raggiungere le famiglie di origine o i genitori separati non vedere i loro figli; ci dite che tanti giovani, uomini, donne, bambini non potranno vivere le festività in famiglia, reclusi nelle Regioni dove lavorano e studiano. Pensate a quanti giovani del Sud sono al Nord a lavorare, che grazie a voi o per colpa vostra non potranno tornare a casa. Ci dite che non potremo spostarci nemmeno tra i Comuni, ci dite che Gesù bambino - perché ormai scrivete anche il Vangelo - dovrà nascere alle 22 anziché alle 24. *(Applausi)*. Ma che differenza c'è tra le 22 e le 24, caro Ministro? Ci dite che non potremo stare in famiglia in più di sei persone e penalizzate le famiglie numerose, perché l'avete detto voi che se ci sono più di sei persone in famiglia non va bene. Ci dite che le scuole Ci dite che le scuole potrebbero aprire prima, l'ho sentito dire anche dai colleghi del MoVimento 5 Stelle. È vero che gli insegnanti vorrebbero insegnare non con la didattica a distanza, ma che cosa avete fatto per tutelarli? [**Presidenza del

dopo che ogni cittadino italiano ha visto quello che è successo a Napoli nei giorni scorsi. Non siete in grado di garantire l'ordine pubblico, non siete in grado di far rispettare le vostre regole. *(Applausi)*. Non siete in grado di permettere ai cittadini italiani di vivere e di avere una vita normale. Ministro, avete fallito, non avete una strategia

finestra") *(M5S)*. Signor Ministro, Governo, onorevoli colleghi, voglio iniziare ponendo l'accento su alcune criticità emerse durante questi mesi di pandemia. innanzitutto doveroso rilevare la disparità e le diseguaglianze nell'applicazione dei provvedimenti adottati dal Governo centrale su tutto il territorio nazionale. Purtroppo la riforma del Titolo V della Costituzione ci ha portati ad avere tanti sistemi sanitari regionali differenti, un modello che ha mostrato tutti i suoi limiti e su cui sarà necessaria una profonda riflessione. Bisognerà seriamente ripensare la gestione sanitaria con l'obiettivo di limitare le sperequazioni esistenti tra le diverse Regioni, che questa pandemia ha semplicemente accentuato, tutto ciò anche attraverso una modifica radicale del Titolo V, condivisa il più possibile da tutte le forze politiche. In molte Regioni, nonostante le risorse stanziate dal Governo, ci sono stati gravi ritardi sia nell'attivazione delle USCA sia nell'aumento del numero dei posti letto di terapia intensiva. In questo senso, per esempio, abbiamo assistito anche a situazioni poco chiare. Nella mia Regione, la Campania, c'è stata confusione con l'utilizzo della formula *escamotage* «posti attivi» come se l'emergenza o l'urgente disponibilità di posti letto potesse essere procrastinata o differita nel tempo e non essere invece un'urgenza immediata, capace di fare la differenza tra la vita e la morte. Altresì, mi premeva evidenziare, signor Ministro, la grossa problematica della medicina territoriale. Durante questa pandemia sono emerse, come sostenuto da tempo dal Movimento 5 Stelle, la necessità di una sua più razionale organizzazione e l'esigenza di mettere in atto un potenziamento - mi lasci dire - indispensabile, signor Ministro, dell'assistenza domiciliare, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione e un più attivo coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. È quanto mai necessario mettere i medici nelle condizioni migliori per poter operare in piena sicurezza per se stessi e i propri pazienti. Allo stesso modo, non sfugge che i medici di base, vere sentinelle e baluardo sul territorio, ricoprono un ruolo fondamentale nella nostra organizzazione sanitaria e che, di conseguenza, occorre che essi acquistino sempre più coscienza del loro ruolo. Servirà potenziare un approccio continuativo e diretto e sempre meno telefonico con i loro pazienti, che in tal modo si sentiranno più sicuri e meno abbandonati, per arrivare, come già detto, alle USCA, attivate in modo disomogeneo e insufficiente in alcune Regioni, come ad esempio la Campania che, secondo gli ultimi dati, ne avrebbe attivate poco più del 15 per cento. La conseguenza logica e drammatica di ciò è costituita dai gravissimi ritardi verificatesi, come segnalato da tantissimi cittadini, sia nell'esecuzione di tamponi ai contatti dei soggetti positivi sia nell'assistenza e nella corretta gestione domiciliare dei pazienti con Covid-19 le cui condizioni cliniche, se monitorate e controllate periodicamente con le opportune terapie domiciliari e secondo i protocolli stabiliti, non necessitano del ricovero ospedaliero, da riservare ai casi più gravi. Sappiamo benissimo che solo l'implementazione di un'adeguata assistenza domiciliare può realmente alleggerire il carico delle strutture ospedaliere. Se analizziamo la problematica Covid, tutti noi diciamo che il virus si diffonde velocemente e l'andamento della curva epidemiologica si modifica rapidamente e continuamente. La conseguenza logica di ciò è che le risposte e tutte le misure adottate devono essere necessariamente commisurate alle varie criticità che via via emergono e modulate per meglio contrastarle e risolverle. Arriviamo a oggi. Tutte le misure individuali e collettive, insieme al senso di responsabilità dei cittadini, rallentano i contagi e la trasmissione del virus. Tuttavia, solo la disponibilità e l'ampia diffusione dell'utilizzo di un vaccino sicuro ed efficace, la sua corretta distribuzione a fasce via via sempre più ampie della popolazione, rappresentano l'arma in più, capace di mettere un punto fermo e decisivo in questa difficile battaglia che il mondo intero sta combattendo, permettendo davvero di tirare un sospiro di sollievo. Da questo momento, con il vaccino, non dovremo sempre inseguire il virus, ma avremo la possibilità di prevenire l'impatto del Covid-19 sul singolo e sulla collettività. L'obiettivo del piano nazionale di vaccinazione anti-Covid sarà quello di immunizzare in tempi ragionevoli circa il 70 per cento della popolazione italiana, ovvero circa 40 milioni di persone. Si tratta di un obiettivo importante, ma non utopistico e una *conditio sine qua* *non* per raggiungere una vera immunità di gregge. È chiaro che per fare questo serviranno l'impegno di tutte le forze in campo e un'operazione scaglionata nei mesi. Sarà fondamentale il confronto con le Regioni per organizzare al meglio una distribuzione attenta e sicura delle dosi di vaccino, il controllo della conservazione delle fiale e la programmazione dei soggetti da vaccinare e delle priorità da rispettare. L'efficacia protettiva dei vaccini anti-Covid al momento disponibili è riconosciuta dalla comunità scientifica, anche se ciascuno di essi ha percentuali diverse di immunizzazione. Aspetti da verificare saranno la durata protettiva nel tempo degli anticorpi indotti e la necessità nel corso degli anni successivi di dosi di richiamo dopo le prime due iniziali. Certo è che, di fronte alle tante immagini di sofferenza e morte, occorreva una risposta che fosse veloce ed efficace ma anche sicura. Sarà importante una corretta ed efficace campagna di informazione, comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini per spiegare l'importanza della vaccinazione e favorirne il più possibile l'adesione volontaria, convinta e partecipata. La campagna vaccinale dovrà dare un messaggio chiaro in merito alla sicurezza dei vaccini, da un lato, ma, dall'altro, dovrà insistere sul concetto che la protezione del singolo è indispensabile anche per proteggere gli altri. Questa campagna deve essere avviata e motivata su scelte consapevoli, ma non obbligatorie. Essere vaccinati è un diritto di tutti, dare a tutti la possibilità di farlo in sicurezza e gratuitamente è un dovere delle istituzioni. Nell'applicazione del piano sarà poi importante il coinvolgimento della medicina di base, non solo per preparare un terreno fertile sul territorio di propensione e disponibilità a vaccinarsi, ma anche per segnalare i soggetti che, per patologia o per età, sono destinati *in primis* a ricevere le dosi iniziali del vaccino. Particolare attenzione sarà rivolta alle RSA al personale che vi opera e ai loro ospiti; attenzione che ritengo fondamentale, considerando il triste sacrificio di vite umane che hanno dovuto subire per il diffondersi della pandemia. Senza dubbio gli operatori sanitari dovranno essere tra i primi a ricevere il vaccino per la loro tutela personale e per la tutela delle persone che assistono. Sarebbe bello, signor Ministro, se tra le priorità venissero inseriti anche i *caregiver* e i genitori con figli con disabilità per il difficile compito di assistenza che svolgono nei confronti delle persone fragili. Questo vaccino rappresenta una speranza e il compito più importante che avremo nei prossimi mesi sarà quello di monitorarne la distribuzione e la somministrazione. Avendo stipulato due grandi accordi con aziende farmaceutiche diverse, Pfizer e AstraZeneca, il nostro Paese avrà sia una maggiore disponibilità di dosi di vaccino sia una tempistica migliore nell'approvvigionamento. Il Governo sta continuando a sostenere le categorie in difficoltà a causa delle chiusure, nella consapevolezza che nessuno deve essere lasciato indietro e che, purtroppo, fin quando non inizierà la distribuzione del vaccino, ma anche oltre, la tutela delle vite umane passerà attraverso l'uso delle mascherine e del distanziamento sociale. Solo così, e concludo, signor Presidente, si potrà ritornare alla tanto desiderata normalizzazione della nostra vita sociale, anche se nulla potrà più essere come prima.

però è bene precisare che la regia del Governo e l'encomiabile lavoro di tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e operatori sociosanitari, sono stati organizzati in tempi brevissimi. Nello stesso tempo, l'operato del Governo e degli operatori sanitari ha permesso un adeguato approccio al grande problema pandemico.

e in particolare con il cosiddetto decreto rilancio, è stato messo in evidenza il ruolo fondamentale della medicina territoriale. È stato altresì ben evidenziato il ruolo del medico di famiglia

il concetto di attività ospedale-centrica deve essere modificato, bisogna intervenire sulla medicina territoriale per i vari motivi che sono emersi emersi durante la fase pandemica. Il paziente deve ricorrere alla struttura ospedaliera solo quando le condizioni cliniche richiedono un'assistenza multispecialistica che a domicilio non è possibile assicurare. Vanno bene quindi i provvedimenti rispettando tutti i comportamenti necessari che ormai tutti conoscono (il distanziamento, il lavaggio delle mani e l'uso della mascherina sono fondamentali), la cosa fondamentale è però, come ha detto il Ministro, l'arrivo del vaccino. Il vaccino è una condizione fondamentale perché si possa determinare l'immunità di gregge,

che una persona su sei non vuole farlo, quindi bisogna dimostrare in tutti i modi e informare che la vaccinazione è fondamentale e dunque mettere in atto un'adeguata campagna informativa.

mi sono soffermato sull'apertura della sua relazione in cui lei ha fatto riferimento alla nostra Costituzione e ai valori e ai valori che essa richiama. Quando a volte si affrontano delle difficoltà sono io il primo, nelle normali esperienze di vita, a fare riferimento ai principi. stiamo certamente attraversando un periodo unico della storia dell'umanità: in un mondo globalizzato, questo invisibile nemico dell'umanità ha raggiunto tutte le parti del mondo. Non è come una volta

questo fenomeno ha pervaso il mondo.

le persone più vulnerabili, le persone anziane e anche qualcuno più giovane che magari non è in buono stato di salute. In questo contesto ritengo allora che non sia assolutamente degno di lode

lanciare questo messaggio alla popolazione. A nessuno può far piacere di essere rinchiuso in casa, però sappiamo che dobbiamo farlo. con un riferimento anche a un fatto personale. Io ci sono cascato in questo problema, ho potuto ricostruire anche i contatti che avevo avuto e per questo sono assolutamente convinto che qualche cautela serve e dobbiamo saperlo comunicare alla popolazione intera, perché l'Italia sta facendo bene e il Governo sta operando nel migliore dei modi possibili.

nella sua relazione il Ministro ha già indicato chiaramente gli assi su cui il nostro Paese si muoverà per quanto riguarda il piano vaccini.

In questi giorni abbiamo promosso, insieme a tanti scienziati e colleghi, un appello, che ha raggiunto e superato le 50.000 firme, per far sì che le parole d'ordine siano «garantire l'accesso universale ai vaccini», l'accesso cittadini ai vaccini. L'auspicio è che queste bellissime parole d'ordine possano effettivamente realizzarsi, perché sappiamo perfettamente che in tutte le pandemie, ma mai come in questa, vi è un problema vero di accesso ai prodotti essenziali da parte di vari Paesi. Ci sono i Paesi più ricchi e i Paesi più poveri, ma anche all'interno dei Paesi più ricchi vi sono grandi disuguaglianze. È un problema che il mondo ha dovuto affrontare varie volte; l'abbiamo dovuto affrontare con l'HIV e con altri virus ed epidemie pericolose.

dei brevetti. Questa è l'unica possibilità (insieme a tante altre ovviamente, ma questa è condizione assolutamente indispensabile) per far sì che l'accesso ai vaccini sia garantito a tutti. Questo riguarda sia i Paesi

Sudafrica e l'India si sono già messi in campo per chiedere a tutti i Paesi dell'Organizzazione mondiale del commercio una deroga rispetto agli obblighi contenuti nell'accordo TRIPS.

dai senatori Romeo, Bernini e Ciriani, e n. 2, dai senatori Pirro, Boldrini, Errani e Sbrollini. I testi sono in distribuzione. Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Signor Presidente, ringrazio tutti i senatori che hanno preso parte a questo dibattito, che è stato senz'altro ricco e potrà aiutarci nel lavoro delle prossime ore. Proverò a replicare brevemente, vista la lunga introduzione che ho voluto fare, ma i temi sono stati tanti, perché, come noto, abbiamo diviso la discussione su due questioni fondamentali: la prima, il prossimo DPCM e il quadro epidemiologico del Paese; la seconda, la presentazione del piano strategico sul vaccino Covid, tema assolutamente prioritario, come noto, per il futuro della nostra comunità. Sul primo punto, in riferimento al piano epidemiologico, dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire con nettezza alla nostra opinione pubblica e a noi stessi che ci sono due verità due verità che possono apparire in contraddizione, ma che in realtà non lo sono. La prima verità è che, da qualche settimana, finalmente, vediamo dati incoraggianti, che segnalano un progresso che va nella direzione giusta. Ho avuto modo di indicare che cosa è avvenuto sul famoso indice di trasmissione del contagio, l'RT, nelle ultime quattro settimane: siamo passati da 1,7 a 1,4, poi a 1,18 e, dall'ultima rilevazione, a 1,08. Questo significa che le misure stanno funzionando e che, un po' alla volta, l'operazione di provare a mettere la curva sotto controllo sta dando i risultati che ci aspettavamo. Questa è una verità con la quale dobbiamo fare i conti,

possano darci ulteriori elementi nei prossimi giorni che vadano ancora nella direzione di una riduzione del contagio, di una riduzione delle persone malate. Se questa è una verità importante che ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, che finalmente c'è una tendenza che ci porta nella direzione giusta, l'altra verità è che c'è ancora una situazione molto complicata nel nostro Paese. I contagi sono, in numeri assoluti, molto elevati; i decessi sono, purtroppo, in numero molto elevato, e ancora la stessa pressione sui posti letto in terapia intensiva e subintensiva e in area medica è molto elevata. Questo ci chiede un approccio di grande cautela e di grande precauzione che dobbiamo considerare indispensabile se vogliamo tenere la curva sotto controllo. Dico un dato su tutti, che mi pare di particolare importanza: ad oggi nel nostro paese ci sono più di 320 casi ogni 100.000 abitanti; è un numero molto alto. Tutti i migliori studi scientifici dei nostri tecnici segnalano come la cifra per riportare sotto controllo in modo particolare il *contact tracing*, il tracciamento, sia quella di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Significa che abbiamo fatto un pezzetto di strada, ma che ancora non basta; dobbiamo continuare a fare un lavoro insistente che ci consenta di riportare pienamente la curva sotto controllo. Per questo abbiamo bisogno, nel prossimo DPCM, di mantenere una linea di rigore, di serietà e di grande cautela e prudenza rispetto a quanto può avvenire. Lo dico in modo particolare rispetto alla peculiarità della fase e della stagione verso cui stiamo andando, e cioè la fase delle festività natalizie, che di per sé porta il rischio di un aumento degli spostamenti, di un aumento dei contatti tra le persone, e che quindi richiede un livello di attenzione ancora più alto. Nel prossimo DPCM l'intenzione del Governo sarà prima di tutto di riconfermare l'impianto a tre colori, con fasce rosse, arancioni e gialle, che ha creato finora le condizioni per rimettere sotto controllo l'epidemia nel nostro Paese. La soluzione che abbiamo messo in campo nel mese scorso con la costruzione di questo impianto per fasce, che dipendono dalla situazione epidemiologica di ciascuna Regione, ha portato un risultato che va nella direzione giusta, quindi dobbiamo confermare questo modello, dietro cui c'è il tentativo - che io ritengo di grandissima importanza - di piegare la curva senza un *lockdown* generalizzato. Questa è la grande differenza con il mese di marzo. Nel mese di marzo, l'Italia è stato il primo Paese a piegare la curva, indicando la strada di un *lockdown* generalizzato. Invece, in questa seconda ondata, stiamo provando a piegare la curva con un modello diverso, che ci consenta di leggere ciò che avviene, territorio per territorio, Regione per Regione, per riportare sotto controllo la curva del contagio, senza farci pagare il prezzo sociale, economico e finanche culturale di una chiusura generalizzata. Il secondo asse del DPCM avrà a che fare con la necessità di gestire, nel modo più accorto possibile, le giornate delle festività natalizie. Proveremo a lavorare per limitare gli spostamenti a partire da quelli internazionali, per limitare gli spostamenti tra le Regioni e, nei giorni più delicati, anche per limitare gli spostamenti tra i Comuni. Dobbiamo evitare in tutti i modi che ci sia una coincidenza, alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio, tra una potenziale fase di recrudescenza del virus e l'avvio di questa operazione

vorrei ribadire l'idea e i principi di fondo, che ci guideranno rispetto alla campagna di vaccinazione per il Covid. Ho sempre detto, dall'inizio di questa epidemia, che sarebbe stata la scienza a portarci fuori da questa battaglia, così difficile e drammatica. La scienza, effettivamente, ci sta consegnando i primi risultati incoraggianti, che devono farci dire, ancora con più forza, forza, che gli investimenti pubblici e privati sulla ricerca scientifica e sui nostri scienziati hanno bisogno di essere rafforzati sempre di più, perché dalla scienza possono venire le soluzioni che tutti aspettiamo.

approvazioni di natura formale, ma abbiamo due date segnate in rosso sul nostro calendario: la data del 29 dicembre e quella del 12 gennaio. In queste due date sono previste le prime validazioni e le prime certificazioni, che dovrebbero arrivare, rispettivamente, per il vaccino Pfizer BioNtech e per il vaccino Moderna. Chiaramente parlo ancora con cautela e con prudenza, perché noi stessi pretendiamo che l'EMA svolga tutti i controlli, tenendo altissima l'asticella della sorveglianza, perché quando un vaccino arriverà

di una cifra molto significativa. Le primissime dosi arriveranno, secondo i nostri auspici e le valutazioni dei nostri tecnici, alla fine di gennaio e poi, gradualmente, si arriverà ad una vaccinazione più ampia, con i momenti fondamentali per la fine della primavera e l'estate. Penso che la scelta più delicata, che oggi ho provato a illustrare al nostro Parlamento, sia quella relativa alle prime categorie che decideremo di vaccinare. Infatti il vaccino arriverà, ma non arriverà subito in tutte le dosi e quindi, nelle primissime settimane, dovremo selezionare le categorie a cui somministrare dette dosi. La valutazione del Governo è di partire dalle categorie più a rischio e più di frontiera, la prima delle quali è sicuramente quella del personale sanitario: i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri professionisti sanitari, che in questa battaglia con il Covid sono sempre stati la prima linea. Vaccinare loro significa rafforzare la resilienza del nostro Servizio sanitario nazionale nonché evitare che un loro eventuale contagio possa trasferirsi ai pazienti, che sono molto spesso portatori di fragilità e quindi più deboli e più a rischio rispetto agli esiti del Covid.

in più in generale, l'altra grande categoria sarà quella degli anziani. Penso che sulla partita della vaccinazione il nostro Paese deve giocare una grande sfida unitaria e mettere in campo tutte le energie di cui dispone. Stiamo parlando della più grande operazione di vaccinazione di massa che si sia mai vista nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di mettere a sistema tutte le energie di cui disponiamo, dalle istituzioni repubblicane, le Regioni, il Governo nazionale, alle risorse alle risorse delle nostre Forze armate e della Protezione civile. Metteremo in campo tutte le energie perché questa è una grande sfida nazionale. È una sfida di tutti su cui dobbiamo assolutamente impegnare ogni energia. Infine, mi sia consentito ribadire che proprio per il senso di questa sfida, noi dovremmo, come Parlamento, unitariamente e senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, dare a tutti un messaggio molto forte di una campagna vaccinale che è la vera grande opportunità per il Paese per provare a superare la fase di difficoltà. Sulla base delle brevi valutazioni

Lo ribadisco perché sulla campagna vaccinale non dobbiamo dividerci per la politica. È un grande obiettivo di tutto il Paese, dunque il mio parere è favorevole sull'impegno

vada nella direzione giusta perché su questa battaglia, su questa sfida enorme di vaccinare milioni e milioni di Italiani ci giochiamo una grande partita come Paese e di tutto abbiamo bisogno tranne che di inutili divisioni.

Signor Presidente, signor Ministro,

Il testo sul quale il Ministro si è espresso è la risoluzione n. 2 a firma Pirro, Boldrini, Errani e Sbrollini che è un testo 1, se è questo che voleva sapere,

Signor Presidente, signor Ministro, anzitutto faccio una precisazione: io e i colleghi Bressa, Cattaneo ed altri voteremo risoluzione della maggioranza, ma, poiché parlo a nome del Gruppo Per le Autonomie, ho l'obbligo morale di spiegare che i senatori Steger, Durnwalder e Laniece non se la sentono di votare la risoluzione della maggioranza per questioni connesse a valutazioni diverse sul tema della montagna, rappresentano territori come la Provincia di Bolzano e la Val d'Aosta e ritengono di avere una posizione critica rispetto ai ai provvedimenti che il Governo ha in cantiere sui temi della montagna e della stagione sciistica. Detto questo, voglio essere brevissimo e dire che in questo Parlamento si sta, come al solito, leggendo lo stesso copione: ci stiamo dividendo tra trionfalisti e disfattisti. I trionfalisti sono pronti a spiegare che il Governo sta sostanzialmente mettendo in campo una sorta di modello che gli altri sarebbero impegnati a copiare, e i disfattisti sono impegnati a spiegare che il Governo ha sbagliato tutto e che in Italia si verifica ciò che non si verifica in nessun'altra parte del mondo. Colleghi, direi di tenere i bollenti spiriti negli armadi, perché non è il caso di scomodare né il trionfalismo né il disfattismo, perché sono entrambi atteggiamenti sbagliati, che peraltro contrastano con una cosa seria che il Ministro ha detto: ha fatto un appello all'unità del Paese per affrontare la tempesta che stiamo vivendo. Vorrei mettere in fila alcune questioni. La prima è la seguente: oggi il professor Cassese sul «Corriere della Sera» - il professor Cassese non è l'ultimo arrivato in Italia, perché non è stato solo membro autorevole della Corte costituzionale, ma è uno scienziato del diritto che tutto il mondo ci invidia - sostiene che abbiamo affrontato una babele istituzionale nel rapporto tra Stato e Regioni. Sono totalmente d'accordo con lui e credo che se ci fosse ancora qualche dubbio, questa vicenda ha confermato la necessità di intervenire legislativamente per chiarire i vuoti che esistono nella nostra normativa e nelle nostre leggi nel rapporto tra Stato centrale e Regioni. Un po' tutti, lo Stato e le Regioni, al reciproco scaricabarile in questa vicenda, salvo poi criticare l'uno o l'altro quando i provvedimenti venivano presi in una sorta di gioco a rimpiattino. Questo è un problema istituzionale e riguarda il centrosinistra e il centrodestra, chi governa oggi e chi governerà domani, perché i Governi passano ma le istituzioni rimangono, e il Parlamento rimane. Credo che questo monito non vada lasciato cadere.

stimati da tutti in questa sede al di là delle visioni, che rischiamo di avere anche una Babele nello Stato. Quando sento ad esempio che, in ordine al *recovery fund* e al tema del MES, sono in gestazione decine di commissioni con centinaia di esperti, ho il dubbio che sia in atto una sorta di commissariamento dei Ministeri. Non credo sia giusto deresponsabilizzare i Ministeri; se i Ministri non funzionano, cambiamo i Ministri, ma non possiamo sostanzialmente una sorta di confusione istituzionale per cui, tra scienziati, commissioni, esperti e Ministri, non si capisce più niente.

e magari, nella confusione di responsabilità, si producono poi soluzioni che, secondo me, non sono le migliori. Vorrei dire una cosa che riguarda due categorie di cittadini del Paese: gli anziani e i giovani. Gli anziani hanno bisogno che venga rispettato il loro bisogno di affettività: la solitudine degli anziani è una delle grandi questioni che la pandemia pone nella sua crudeltà.

sono profondamente frustrati, perché i nostri figli, di 12, 13, 15 o 16 anni, vivono per la loro socialità scolastica e hanno la necessità che la scuola sia aperta a tutti i costi. Certo,

perché, se poi si accalcano sui trasporti...

credo che le dispute ideologiche sul MES non servano, così come ritengo sia necessario utilizzare questo strumento per adeguare un sistema sanitario che, soprattutto negli aspetti di prevenzione di base, ha grandissime lacune.

se riusciremo ad agganciarci al vaccino - lei ci ha detto che a gennaio probabilmente riusciremo a fare già le prime vaccinazioni su circa 1.700.000

estate. L'altro treno da agganciare è quello del *recovery*. Infatti, una volta chiusa la vicenda dell'emergenza sanitaria (speriamo presto), avremo da fronteggiare una crisi economica che per ora stiamo anestetizzando grazie ai ristori e agli interventi che lo Stato sta facendo in maniera straordinaria proprio per le perdite economiche, ma che esploderà

eventualmente questa campagna di vaccinazione non dovesse avere gli effetti sperati, si potrà procedere con l'obbligo vaccinale. va bene così, l'importante è che l'obiettivo sia l'immunità di gregge perché non vorremmo sostituire le categorie oggi a rischio (le persone più anziane

di persone immunodepresse e malati oncologici che non possono vaccinarsi e hanno bisogno dell'immunità di gregge per poter sopravvivere. Pertanto, dobbiamo evitare di scambiare soltanto chi è a rischio; dobbiamo risolverlo definitivamente questo problema. L'immunità di gregge sarà indispensabile. Ugualmente indispensabile è contrastare una campagna «No Vax» veramente invasiva e pesante. Spesso accade che parte della politica e dei partiti politici strizzino l'occhio a questi No Vax con le modalità

su alcuni milioni di cittadini e sul potenziamento di un vaccino a cui comunque siamo abituati, abbiamo riscontrato delle difficoltà. Quando dovremo fare una campagna di vaccinazione che dovrà riguardare almeno 40 milioni di persone in tempi brevissimi, queste difficoltà si potrebbero amplificare

ci affidiamo soltanto alle ASL, ai medici di base e a chi ha dato una mano nel periodo del vaccino antinfluenzale, di fronte ai milioni di vaccini da fare, rischiamo di trovarci in difficoltà. È importante non sbagliare.

delle lezioni per non commetterli un'altra volta perché il passaggio del vaccino è decisivo e non ci possiamo permettere assolutamente di sbagliare. Pertanto, va bene il piano che lei ci ha sottoposto. Ministro, sento sempre il disco rotto di chi dice che dobbiamo andare a casa, che non siamo in grado, di chi dice: «Ci vogliono rubare il Natale». Questa è stata l'espressione che ha utilizzato Salvini parecchie volte.

mettere in sicurezza sanitaria il Paese è la nostra priorità. Dobbiamo superare l'ultimo miglio con l'Epifania, con l'ultimo giorno di ipotetiche feste natalizie. Dopodiché potremo finalmente far ripartire il Paese.

sono state le stesse persone che, quando siamo ripartiti e c'era l'effetto dell'ondata estiva, ci hanno chiesto dove fosse il Governo quest'estate; sono le stesse persone che ora ci dicono: «Perché dovete chiudere a Natale? Facciamo festeggiare il Natale»; poi saranno gli stessi che ci diranno: «Per quale ragione avete riaperto a Natale, visto che c'è un'altra ondata?».

è chiaro che sarà sempre questo l'atteggiamento. Pertanto, ascoltiamo le idee migliori, ma, al tempo stesso, stiamo lontani dalle strumentalizzazioni.

quindi continuare a insistere su uno strumento che sta funzionando. Tutti quelli che hanno stigmatizzato le Regioni colorate di giallo o di rosso e che ci prendevano in giro dovrebbero ricredersi rispetto all'efficacia dell'azione messa in campo. Naturalmente, signor Ministro, noi dobbiamo avere avere molto rispetto dei passaggi sacri che si tengono in Parlamento. Quando si decide di anticipare provvedimenti del Governo sul tema

quella dei trasporti e quella dell'istruzione, perché l'una parla per l'altra, mentre noi vorremmo che ognuna delle due parlasse del suo settore di competenza. Si coordinassero, parlassero un po' meno e facessero un po' di più, perché questo è un tema assolutamente delicato. *(Applausi)*. Non capiamo altresì perché si debbano impedire, ad esempio, le crociere, che sono luoghi in cui possono essere fatti i tamponi per tutti e sono tutti sotto controllo.

perché l'abbiamo detto e fatto fino ad ora, non sempre prontamente, ma gli ultimi ristori sono andati molto bene e dobbiamo garantirli anche successivamente.

è quella dedicata alla piaggeria e l'ultima è quella riservata alle cose che non vanno. Se allarghiamo l'ultima parte e riduciamo la prima, forse riusciamo a combinare qualcosa di buono.

e invece ci ha relazionato per due terzi del suo intervento sul tema dei vaccini. Va benissimo, naturalmente, e la ringraziamo per quanto ci ha detto, ma rimangono alcuni passaggi, su questo tema, che ci preoccupano fortemente. Il primo è che affidiamo la parte distributiva, cioè la logistica, cioè la gestione di un intero piano vaccinale,

non aspetta altro che qualcun altro faccia il suo lavoro, visto che lui apertamente ha dichiarato, ad esempio, che la *app* Immuni ha fallito e, avendola fatta lui, è una sorta di reo confesso in una chiamata in correità rispetto al Governo.

Benissimo, ben fatto, ma vorrei farle osservare, Ministro, che nel Regno Unito cominciano a vaccinare la settimana prossima. cominciano a vaccinare la settimana prossima. Mi perdoni, Ministro, ma come giudico la bontà di un'operazione fatta dal Governo se non con la rapidità? Questo è un problema tempo-dipendente, come l'infarto. inglesi vaccinano la settimana prossima e noi vacciniamo a primavera, come lei ha detto, signor Ministro, non so se si è reso conto di questo passaggio. Lei ha detto che la gran parte del nostro piano vaccinale si esplicherà a primavera. Noi vaccineremo, con quanti mesi di ritardo rispetto ad altri Paesi che non hanno seguito il percorso nell'ambito delle istituzioni europee? Lei si è vantato di non aver utilizzato quella clausola che ci dava modo di fare l'una e l'altra si è vantato del fatto di non aver agito andando oltre il sistema messo in campo dalle istituzioni europee e invece avrebbe dovuto semplicemente aprire i due canali, in modo da poter usufruire di quello che prima ci dava modo di cominciare a vaccinare. Un'altra questione su cui lei ha taciuto, Ministro, mi perdoni, è quella riguardante il piano pandemico nazionale. È su tutti i giornali, è sulla bocca di tutti, lei non può tacere su queste circostanze. È venuto in Parlamento e qualcosa rispetto alle dichiarazioni di Ranieri Guerra ci dovrebbe dire

signor Ministro, dichiara che il piano che noi abbiamo a disposizione è privo della data di pubblicazione e di alcuna bibliografia, il che ha consentito di spacciarlo più volte come nuovo

non viene delineata una chiara struttura di coordinamento, comando e controllo, come è invece riportato in tutti i piani degli altri Paesi. L'assenza di un piano pandemico nazionale è la fonte di tutti i problemi che abbiamo riscontrato in questi mesi.

al *treating*, abbiamo denunciato l'assenza di protocolli di trattamento. Il protocollo tirato fuori solo qualche giorno fa non contiene le indicazioni utili e indispensabili, ossia il ai farmaci. I medici di medicina generale non hanno protocolli per la continuità assistenziale e le cure domiciliari e in ospedale c'è un mare di inappropriatezza sia in ingresso, che in uscita.

se lei gioca a tressette, questo funziona quando si gioca una carta e si dice come passa. Ma noi siamo - o dovremmo essere - legislatori e, in un momento di grave emergenza come questa,

come vivere il Natale e non ce lo deve venire a dire il presidente Conte in televisione a beneficio di telecamera. Signor Ministro, basta con apparizioni in televisione di gente come il sottosegretario Zampa. Io salvo Sileri perché almeno si attiene ai fatti e, per questo, gli faccio un minimo di

Mi perdoni, però, come farà ad essere obbligatorio il vaccino? Cosa vi inventerete? Lei ha detto che state valutando l'obbligatorietà dei vaccini. Come farete?

infatti sono fallite l'App immuni e l'indagine sierologica, se non avete attuato tutto quello che le Camere vi avevano suggerito, compreso questo ramo del Parlamento con una

Allora spostiamo il Natale, spostiamolo di due ore. Faccio una proposta: allunghiamo di un paio di mesi, visto che la campagna vaccinale parte a primavera, accorpiamolo al 25 aprile e al primo maggio così abbiamo fatto contenti tutti, fanfara festa

ma non basta più l'atteggiamento, che io più volte le ho descritto che è quello del democristiano. Fra l'altro, è presente il presidente Casini che su questo la batte e - diciamo Faccia il suo compito, eserciti il suo ruolo, ma lo faccia con decisioni chiare agli italiani, alle istituzioni

Cercando di fare un ragionamento un po' diverso da quelli che ho ascoltato fino ad ora, vorrei provare a proporre a tutti noi

Partiamo da un dato; credo onestamente possa essere riconosciuto zonizzazione che abbiamo fatto, essa abbia dato esiti positivi. Si è ridotto l'indice Rt e molte Regioni hanno raggiunto un risultato importante. Siamo fuori dal tunnel? No e a questo proposito io spero (e sono sicuro che il Governo lo farà) che l'esperienza dell'estate sia un'indicazione e un monito per tutti noi. Spesso accade che quando si assume la decisione di restringere un'attività piuttosto che un'altra, si discuta e si intervenga per dire che deve essere aperta e che, viceversa, quando ciò non accade si chieda di chiudere. Questo è accaduto, colleghe e colleghi, a tutti in tutti questi mesi.

evitando - faccio un appello - la discussione e le contrapposizioni che ci sono state in queste settimane. hanno bisogno di chiarezza, hanno bisogno di capire le finalità delle scelte in modo trasparente e credo che il Governo sarà pienamente in grado di farlo.

cioè, la norma, non basta il DPCM, non basta la delibera del Presidente; occorre un clima, una condivisione complessiva che riesca a fare in modo che questo periodo importante dal punto di vista familiare, degli affetti, delle relazioni, non non possa replicare ciò che è accaduto nell'estate che ci sta alle spalle. Questo è importantissimo, perfino di più della norma specifica su questo o quell'intervento.

Dato che uno dei temi di questa vicenda nasce dal fatto che il Parlamento non ha mai desunto i principi fondamentali dell'articolo 117 della Costituzione, facciamo la riforma della sanità e in quella desumiamo i principi fondamentali, perché il sistema sanitario è nazionale

non sia il caso di dargli una forza legislativa di norma primaria, in modo tale che sia chiaro a tutto il Paese, a tutti i soggetti interessati alla sua gestione, che il piano si applica interamente, su tutto il territorio nazionale, in modo è una scelta positiva importante, anzi un lavoro importante che è stato compiuto a livello europeo per i vaccini.

e globale, per fare in modo che i vaccini anti-Covid vedano il superamento dei brevetti e dei diritti di proprietà. È una scelta strategica che riguarda il mondo e tanti Paesi che diversamente rischierebbero, con conseguenze gravissime, di non potere avere il vaccino. Sulla base di questi principi approviamo le sue comunicazioni e confidiamo in un ruolo e in una forza del Governo nel costruire questo impianto comune della Repubblica.

Affrontare il Natale è un passaggio importante, perché lo facciamo con un carico di consapevolezza maggiore rispetto a nove mesi fa. Abbiamo conosciuto meglio il virus, sappiamo quanto sia pericoloso e sappiamo quanto sia capace di trasmettersi attraverso le persone nei momenti di socialità e di assembramento. Conosciamo l'impatto del virus sul nostro sistema sanitario, sappiamo anche quale sia l'impatto del virus sulla vita sociale di giovani, di famiglie e di anziani e conosciamo le ricadute sul sistema economico e delle imprese del nostro Paese, specie quelle degli esercizi pubblici e del turismo. Ma sappiamo anche quale sia l'efficacia delle azioni di contrasto alla diffusione del virus, perché abbiamo sperimentato differenti intensità di provvedimenti, sempre con l'obiettivo di salvaguardare la salute e poi di contenere tutti gli altri effetti negativi sulla comunità e sull'economia. Ad una prima risposta alla pandemia, cioè il *lockdown* nazionale generalizzato attuato in primavera, che non ha eradicato il virus, ma non poteva farlo per evidenti differenze di azione tra gli Stati europei, quando il virus ha ripreso a trasmettersi alla fine dell'estate abbiamo fatto seguire una risposta graduata e differenziata sul territorio nazionale, basata su un sistema di monitoraggio che sta funzionando. La colorazione delle Regioni è il modo sintetico per descrivere sia lo stato di fatto della pandemia, sia le relative indicazioni sui comportamenti da seguire per ridurre i contagi. La sua relazione, signor Ministro, dà atto di questa efficacia e la tendenza ci porta a ritenere che alla vigilia di Natale buona parte delle Regioni saranno in zona gialla. Solo se fosse veramente così, nonostante questa previsione sia realistica, ci appresteremmo a mettere in atto delle azioni che aumenteranno nel periodo natalizio i vincoli proprio delle zone gialle, con impatti molto diversi da Regione a Regione. Conosciamo tutti cosa significa il periodo natalizio in termini di movimentazione di persone e merci e comprendiamo i rischi maggiori che si verifichino situazioni fuori controllo, ma sappiamo anche che se non può essere un "liberi tutti", allo stesso modo non può essere una cortina di ferro. Questo ci deve muovere con l'intento di contenere in modo adeguato e dare maggiore ordine alle attività che a Natale i cittadini e le famiglie si aspettano di poter fare almeno in una certa parte, perché sarà comunque un Natale diverso con dei sacrifici da affrontare. Oggi si può fissare una linea di rigore, ma questa può reggere soprattutto se quando la comunichiamo si rafforza nei cittadini la convinzione che i comportamenti responsabili sono la base per la lotta alla pandemia che stiamo conducendo a tutti i livelli istituzionali. Se fissiamo una linea di rigore che non genera convinzione e adesione da parte dei cittadini, rischiamo effetti controproducenti. Proprio per il carico di consapevolezza che ho descritto prima, al netto dei focolai che dovessero manifestarsi, ci si deve orientare comunque su azioni che consentano una coerenza su tutto il territorio nazionale delle misure relative alle aperture delle attività economiche affinché, per esempio, non vi siano zone dove gli alberghi possono stare aperti e zone dove devono restare chiusi. Allo stesso modo, crediamo che siano da prendere in considerazione - per una valutazione più attenta azioni che consentano alle famiglie di ricongiungersi con genitori anziani soli anche tra Regioni diverse e anche in dimore diverse dalla residenza. Il tema delle scuole è decisivo per il futuro del nostro Paese. Vogliamo le scuole aperte in sicurezza, ma ciò significa che possono essere riaperte solo quando tutta la filiera interessata sia in condizioni di sicurezza: dal sistema dei trasporti fino all'organizzazione di eventuali turni di ingresso e svolgimento delle lezioni. Le comunicazioni del ministro Speranza ci mettono in un'attesa che ragionevolmente non andrà delusa riguardo alla disponibilità dei vaccini nei prossimi mesi. Condividiamo gli obiettivi e la strategia del Ministro riguardo alla gestione della distribuzione dei vaccini alla quale ci stiamo preparando. Si tratta delle giuste premesse per la costruzione di un piano operativo che necessita di un dispiegamento di risorse umane e organizzative, che giustamente va gestito in modo centralizzato,

Comprendiamo che per il sistema sanitario si tratta di una sfida nella sfida: gestire il decorso della pandemia nel mentre si affronta la campagna vaccinale. Il coinvolgimento delle Forze armate attraverso l'indirizzo del ministro Guerini sarà decisivo per dare tempestività ed efficacia al piano operativo di vaccinazione. Le Forze armate, una volta di più, si dimostrano un'insostituibile infrastruttura del Paese integrata nei processi di gestione e di superamento delle emergenze. Voglio sottolineare, a questo punto, il lavoro fatto dal ministro Speranza sul piano europeo sia per coordinare le azioni di contenimento della pandemia - e il DPCM relativo al periodo natalizio sarà un passaggio importante di verifica - sia per impostare in modo adeguato la gestione europea di opzione, acquisto e distribuzione dei vaccini. L'iniziativa dell'Italia ha contribuito ad allineare l'Europa su un più alto livello di considerazione da riservare ai sistemi sanitari nazionali. Se così non fosse, non saremmo giunti alla storica proposta di modifica della natura dei fondi MES, susseguente alla modifica delle modalità per il loro utilizzo, ma su questo voglio esprimere una valutazione, e vado a concludere. La nostra discussione nazionale è tutta centrata su quello che deve fare l'Europa. invece, che sia giunto il momento di concentrarci su quello che deve fare l'Italia. Signor Ministro, da settimane abbiamo chiara la necessità di un piano strategico di modernizzazione della sanità italiana che espliciti la visione che vogliamo attuare affinché il sistema sanitario italiano sia in grado di affrontare nuove eventuali sfide pandemiche, ma con la capacità di assicurare la continuità terapeutica e di intervento per le altre patologie. Lei è venuto in quest'Aula e questi discorsi li ha ascoltati molte volte. Abbiamo messo risorse significative per affrontare l'emergenza per le assunzioni, per i Covid *hospital*, ma non abbiamo definito un progetto che chiarisca gli investimenti che cambiano la nostra sanità con servizi territoriali diversamente organizzati, come la telemedicina, con un ridisegno dei ruoli sul territorio, con nuove tecnologie per la prevenzione e la cura. Credo sia giunto il momento di presentare questo progetto e così capiremo tutti a cosa servono all'Italia i 35 miliardi di risorse del MES. Se il progetto degli investimenti che disegnano la sanità di domani non viene prodotto, signor Ministro, potremo discutere ancora sull'Europa, ma la discussione non avrà costrutto. Certo, c'è anche il tema finanziario, perché quest'anno abbiamo contratto 100 miliardi di euro di debito e ne dovremo restituire più di 100. Invece, per quel che riguarda i 35 miliardi di euro del MES, ne dovremo restituire meno di 35. Il progetto che chiarirà la dimensione degli investimenti nella sanità,

di dosi, che dovrebbero essere sufficienti per la doppia vaccinazione, come ha detto il signor Ministro, e per approntare la riserva di alcune scorte.

mettendo insieme tutto, anche quello che non va messo insieme. Il MES sanitario è un'opportunità per il nostro Paese: si tratta di 37 miliardi di euro, che ci servono immediatamente

- è la seconda volta che lo dice - vuole rivedere il sistema della sanità: vedo strisciante uno statalismo, che non ci piace *(Applausi)*. Signor Ministro,

di essere efficace, efficiente, all'avanguardia, con delle attrazioni anche a livello europeo, vista la loro valenza. Non torniamo indietro su queste cose, perché abbiamo già visto cosa vuol dire centralizzare. Manca dunque qualsiasi riferimento

Abbiamo assoluto bisogno di dare certezze, indicazioni e per questo, presidente Casini, ci vuole la politica, quella con la P maiuscola,

che siano necessarie idee più precise rispetto a quelle che ci avete illustrato fino adesso. Ci sembra che sopravanzi un pensiero molto, molto debole dal punto di vista della soluzione delle problematiche attuali. C'è una visione solo contingente che non ci permette di comprendere come porteremo il nostro Paese fuori da queste secche. Siete anche disordinati, ma la nostra economia è forte e comprende eccellenze in molti settori diversi. Abbiamo bisogno di un Governo che metta al centro l'impresa, che metta al centro il lavoro con regole chiare e precise.

Noi riteniamo, signor Ministro, che vi sia una evidente esagerazione nelle restrizioni delle attività economiche. Anziché volare alto, la maggioranza si aggrappa a vecchie e logore bandiere identitarie per dare soddisfazione ai propri tifosi, ai propri fan. Così i 5 Stelle si aggrappano al rifiuto del MES sanitario, LeU e parte del PD propongono una patrimoniale, ma l'ABC insegna che in un momento di crisi economica tassare ulteriormente vorrebbe dire dare il colpo di grazia all'Italia. *(Applausi)*. Dal punto di vista mediatico, un po' di rumore siete riusciti a farlo. È un danno di immagine che fate al nostro Paese.

che anziché individuare un Ministro unico competente, avete fatto una triplice con sotto trecentocinquanta consulenti con tutti i lavori dei Ministeri sottostanti che hanno tirato fuori dagli archivi vecchi progetti stantii e superati. *(Applausi)*. Bisogna semplificare e voi complicate. Attraverso il Next generation EU, l'Italia arriva ad avere 209 miliardi complessivi. Dobbiamo definire il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza entro aprile 2021. Le risorse andranno poi spese entro il 2026. Se non procediamo con linee di semplificazione e non sburocratizziamo, stiamo assolutamente certi che non arriveremo in tempo ad avere tutti gli atti amministrativi necessari per tradurre questi progetti in realtà. Bisogna superare la crisi economica e sociale che è causata dalla pandemia. Va accelerata la trasformazione del nostro Paese in senso moderno. Le categorie sociali si stanno lamentando, signor Ministro.

ma concretamente e realmente. I soldi non arrivano o non sono arrivati tutti. A mezzanotte di domenica si saprà se si devono pagare o meno le tasse. Signor Ministro, siamo in un momento in cui il Paese richiede uno sforzo

proviamo a costruire e a offrire spunti per andare avanti insieme; l'abbiamo dimostrato come centrodestra, senza che nessuno ci dovesse fare lezione: abbiamo votato unitariamente lo scostamento di bilancio, perché finalmente, invece di fare regalini agli amici degli amici, monopattini e banchi con le rotelle, abbiamo deciso di aiutare partite IVA, lavoratori autonomi, professionisti e artigiani. E il centrodestra c'è stato. verifichiamo cosa non ha funzionato, per provare a far meglio nelle prossime settimane. Innanzitutto, faccio una premessa su infermieri e personale sanitario:

È una presa in giro. Se, Dio non voglia, si arriverà allo sciopero generale indetto dai sindacati per il pubblico impiego, perché il Governo non ascolta è una presa in giro per chi sta combattendo oggi negli ospedali contro il virus e per tutto il popolo del lavoro autonomo e del lavoro dipendente privato,

l'una: o hanno qualcosa di sbagliato a Londra o non funziona qualcosa da noi. Abbiamo letto però che l'Agenzia europea del farmaco ha convocato una riunione d'urgenza per entrare nel merito dei vaccini. Badate bene, oggi è il 2 dicembre e la riunione d'urgenza a Bruxelles è stata convocata per il 29 prossimo venturo: c'è un concetto di urgenza che sul pianeta Terra è diverso rispetto al pianeta Europa. Quindi, signor Ministro, mettiamoci d'accordo. In Turchia partono la settimana prossima - questo è il massimo - con il vaccino che arriva dalla Cina. Dovremo prima o poi portare anche in quest'Aula un momento di chiarezza, perché non è possibile che il Paese che ha contagiato il resto del mondo poi faccia *business* curando il mondo che ha contagiato. *(Applausi).* Qualcuno dovrà dare spiegazioni su quello che non è stato fatto a Pechino.

Nei mesi della pandemia - lo dico per chi ci segue da casa, perché chi è in questo Palazzo lo sa - al commissario Arcuri sono state affidate: la gestione delle mascherine e dell'ossigeno (pessima); la gestione della riapertura delle scuole (pessima); la gestione dell'*app* Immuni (fallita). Adesso, *ad adiuvandum*, gli è stata affidata la soluzione del problema dell'Ilva di Taranto, il mio pensiero e il mio abbraccio vanno agli operai e ai cittadini di quella città *(Applausi)*, perché, se sono in mano a questo signore, hanno poco di cui stare tranquilli. Visto che ha avuto successo su tutto, gli diamo anche la gestione dei vaccini. Mi risulta - signor ministro Speranza, verifichi se è vero - che le associazioni sindacali del trasporto le associazioni sindacali del trasporto da settimane abbiano dato la loro disponibilità a trovarsi intorno a un tavolo del Governo per organizzare il trasporto e la distribuzione dei vaccini, se e quando arriveranno, ma che nessuno le abbia contattate. Se siamo una Repubblica fondata sul commissario Arcuri e sulle *task force*, cambiate la Costituzione; altrimenti, ascoltate il Paese *(Applausi),* perché, visto com'è andata in passato, rischiamo di fallire in futuro. signor Ministro, che la prossima volta si riesca a parlare con lei anche dei problemi dei milioni di malati non Covid: ci sono liste d'attesa spaventose, visite e operazioni rimandate; c'è il mondo dei malati oncologici, che sono in fila come gli altri e non se lo meritano, mentre lottano contro il cancro, e che qualche disgraziato collega senatore ritiene italiani di serie B.

Ringrazio quei medici che, *sua sponte*, stanno salvando migliaia di vite, così come quei farmacisti che, *sua sponte*, stanno mettendo a disposizione i loro spazi per eseguire i tamponi all'esterno delle farmacie, cosa che è vietata questo è surreale. Fra i 6.000 DPCM che Conte ci ha regalato in questi mesi, non avete trovato il modo di cancellare un Regio decreto del 1934 che vieta ai farmacisti di fare punture e tamponi nelle loro sedi. Nel prossimo DPCM superate almeno quest'eredità del passato e permettete ai farmacisti di fare il loro lavoro.

col cappellino, la trombetta e il trenino sulle note di «Maracaibo» di fantozziana memoria. Nessuno pensa all'urgenza di andare a trovare l'amante o il fidanzatino di sedici anni dall'altra parte d'Italia; però, siccome avete deciso - questo leggiamo sui giornali di chiudere gli italiani in casa e nei confini del loro Comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno, almeno ricordatevi non di chi avrebbe voglia di andare a farsi un giro sulla tavola da *snowboard* sulle montagne italiane, ma dei milioni di genitori separati o divorziati che vivono in Italia e dei loro figli di bambini che hanno diritto, almeno a Natale, di stare con la mamma e con il papà; e, se il papà sta a Milano e la mamma a Palermo, chi bloccherà quel papà o quella mamma? C'è un mondo di genitori separati o divorziati e di nonni che non vedono i nipoti: non stiamo parlando di qualche viziato che vuole andare a divertirsi. *(Applausi)*. Questa è l'Italia,

Mi sembra il modo peggiore di celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, portando ulteriore burocrazia nelle sedi di quel terzo settore e di quel volontariato che in questi mesi hanno fatto miracoli in Italia

non è nato in classe, ma, come tutti avevano previsto, fuori dalle classi. Mi spiega che senso ha chiudere i romani a Roma, i palermitani a Palermo e gli aostani ad Aosta il giorno di Natale e di Santo Stefano e poi far viaggiare migliaia di persone sulla stessa metropolitana, sugli stessi autobus e sugli stessi treni? *(Applausi)*. Forse il contagio in montagna è più pericoloso di quello in città?

e questo i mesi scorsi dovrebbero averlo insegnato - è che al 2 dicembre manca una programmazione. Non è possibile che chiunque abbia un'azienda, un negozio, uno studio professionale o un'attività artigianale il 2 dicembre sappia ancora cosa gli succederà fra 20 giorni. Non è possibile, signor Ministro, navigare a vista di settimana in settimana, con sindaci che non sanno, governatori che non sanno, precari, stagionali, operai e commercianti che non sanno. Una volta che avete preso la decisione, portatela avanti

e di cui peraltro oggi leggiamo sulla prima pagina de «La Verità». Dico ai colleghi che giustamente rivendicano "onestà, onestà, onestà!" che in procura a Roma

c'è qualcosa che non sappiamo, altrimenti non si può parlare di merito e premiare chi non lo riconosce. ministro Speranza, ascolteremo ciò che la comunità scientifica ci suggerirà. Spero che in questi pochi minuti abbia colto il fatto che vogliamo costruire,

agli studenti e ai lavoratori che stanno a mille chilometri da casa e che almeno il giorno di Natale e di Santo Stefano non vorrebbero fare festini o festoni,

sequestrati in Libia, perché il Governo per loro non ha mosso un dito. *(Applausi).* Avete speso milioni per riportare in Italia gente che andava in giro per il mondo a farsi gli affari suoi e non state spendendo una lira per riportare in Italia lavoratori del nostro Paese. *(Commenti).* Buon Natale a tutti!

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei ringraziarla per la puntualità della sua informativa. Siamo tutti purtroppo consapevoli o dovremmo esserlo del momento che ancora oggi stiamo vivendo. Dovrebbe esserlo anche il senatore Centinaio, ma non lo sembra: dovrebbe sapere che il suo *leader* si presentava in Senato senza mascherina dovrebbe sapere che quest'estate hanno organizzato un comizio che si è tramutato in un focolaio; dovrebbe sapere che quest'estate le Regioni guidate dalla Lega non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto e siamo arrivati a settembre con ritardi non certo dovuti a chi aveva stanziato le risorse mesi prima, come ha fatto questo Governo. È vergognoso sentire queste parole in Aula. L'Esecutivo ha sempre dato regole precise, fondate sulla responsabilità e sulla tutela della salute e, se qualche persona non le ha rispettate, è anche grazie al pessimo esempio che ha dato chi siede alla mia sinistra in questo emiciclo.

Non capirlo significa andare contro dati scientifici e non rendersi conto della situazione che sta vivendo tutta l'Europa. protegge evitando cenoni, abbracci, veglioni e, in qualche modo, lo spirito di Natale, che è quello di stare tutti insieme. Purtroppo quest'anno stare insieme è proprio ciò che non possiamo permetterci. Grazie alle misure messe in campo dal Governo e da lei, siamo riusciti a contenere finora questa seconda ondata, che comunque è stata violenta, ha messo nuovamente in difficoltà il nostro Sistema sanitario e ha visto perdere la vita a moltissime persone.

Potrei ricordare che, a causa dei tagli fatti negli anni passati, la nostra medicina territoriale è stata indebolita a tal punto da non riuscire a sostenere le necessità dell'emergenza. Potrei ricordare che, da quando il MoVimento 5 Stelle è al Governo del Paese, abbiamo invertito questa tendenza, arrivando a stanziare oltre 12 miliardi di euro, gli ultimi 4 dei quali con la legge di bilancio di quest'anno. Ancora, potrei ricordare che chi prima di noi non aveva programmato il fabbisogno dei medici specialisti ha fatto sì che ora manchino e che i bandi vadano deserti, altro aspetto su cui il MoVimento 5 Stelle è intervenuto, sia aumentando i contratti di formazione specialistica, sia creando una struttura che programmi proprio in base al reale fabbisogno del Sistema sanitario nazionale. Potrei ricordare che aver dato soldi pubblici ai privati, come ha fatto la Lombardia, si è rivelato un fatale errore

Potrei ricordare che le Regioni che quest'estate hanno permesso la riapertura delle discoteche - alcune anche con modalità rimaste oscure, come in Sardegna - hanno commesso una leggerezza, non controllando a dovere cosa poi vi succedeva. Oggi siamo qui e, anziché parlare degli stabilimenti balneari e delle discoteche, parliamo degli impianti da sci. Sarebbe davvero un errore imperdonabile abbassare la guardia in pieno inverno, con ciò che ne conseguirebbe. Sarebbe un errore imperdonabile non rendersi conto che in questo momento l'unica priorità dev'essere la tutela della salute. Il Governo ha approvato un quarto decreto ristori, che serve proprio a sostenere le imprese in difficoltà e i lavoratori. Pensare di sacrificare vite umane a interessi economici, però, è una scelta che, in tutta coscienza, nessuno può prendere. A gennaio inizieranno ad arrivare i primi vaccini e cominceremo a intravedere la luce in fondo al tunnel. Le nostre vite, nel giro di qualche mese, inizieranno a tornare alla normalità. Per inciso, dovremmo inserire nei protocolli per le quarantene l'esonero per chi ha già contratto il Covid-19 e per chi si vaccina, magari prevedendo a supporto un test sierologico che attesti un adeguato titolo anticorpale. Ma torniamo a noi. Ricordiamoci il prezzo che ha pagato la Lombardia alla richiesta sguaiata di qualcuno: Milano deve ripartire! Non dimentichiamoci il sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari. In oltre 200 hanno perso la vita per aver messo davanti alla propria la cura degli altri. E noi, con tutto il rispetto per gli operatori turistici, siamo convinti che non si possa mettere lo sci davanti alla vita degli operatori sanitari. Le misure che prendiamo oggi sono quelle che servono. Non raccontiamo a imprenditori e lavoratori in sofferenza che si potrebbe fare diversamente. È una speculazione indegna. Ci saranno i ristori e gli aiuti (questo Governo ha stanziato oltre 100 miliardi dall'inizio dell'emergenza) e dopo Natale si tornerà a fare il punto della situazione in corso. Veniamo poi al vero elemento di speranza di cui il Ministro ha parlato oggi: i vaccini. Sono state manifestate alcune perplessità sulla loro sicurezza e per alcuni sono arrivati troppo in fretta. La prima cosa da dire, allora, è che il nostro Servizio sanitario nazionale non metterebbe mai a disposizione un farmaco non ritenuto sicuro. poi il nodo della distribuzione. Signor Ministro, sappiamo che ci sono diversi vaccini, con diverse modalità di conservazione. Ciò che stiamo scongiurando è che questo piano sia applicato con modalità diverse nelle diverse Regioni italiane, come purtroppo abbiamo visto fare fino ad ora per tutte le misure che questo Governo aveva responsabilmente messo in campo. Al di là del Titolo V, che dev'essere assolutamente rivisto, è dunque evidente come adesso sia necessaria una supervisione. Non dobbiamo permettere che ai cittadini del Nord venga garantita una cosa, a quelli del Centro un'altra e a quelli del Sud un'altra ancora. Siamo di fronte a una sfida enorme con questo piano vaccinale: la conservazione, la distribuzione e la somministrazione. A chi prima e a chi dopo verrà stabilito in base a criteri medici e scientifici, ma deve essere scritto su pietra che grazie all'impegno di questo Governo ogni cittadino italiano avrà le stesse opportunità e le stesse tempistiche e soprattutto che tutti potranno accedere al vaccino in modo gratuito. Detto questo, voglio concludere il mio intervento facendo un appello agli italiani: siamo stati travolti da una pandemia, abbiamo reagito e stiamo continuando a reagire. Il Covid-19 non va sottovalutato e nemmeno i suoi rischi, lo abbiamo visto. Questo Governo ha sempre agito con coerenza e lo farà anche per le prossime festività, continuando a sostenere lavoratori e imprese con tutti i fondi necessari lo sapete: è stato appena approvato l'ultimo decreto e parliamo di oltre 18 miliardi). oltre 18 miliardi). Torneremo a stare insieme e ad abbracciarci, ma farlo oggi significherebbe rischiare la salute dei nostri genitori e dei nostri nonni: un rischio che non vale la pena, a dispetto di quello che avete sentito dire da qualche sedicente irresponsabile che nei mesi ha strizzato l'occhio ai negazionisti, salvo poi venire a lamentarsi in quest'Aula dell'aumento dei contagi. *(Applausi)*.

parto dalle sue parole: non bisogna perdere la memoria; la aiuterò. Le confesso che ero curioso di vedere con che faccia si sarebbe presentato dopo le inchieste di «Report», la sua, quella di un Ministro che a luglio ha scritto un libro il cui titolo, «Perché guariremo», la getta nel ridicolo. Complimenti: è l'unico autore che riesce a farsi stampare un libro perché non sia venduto. A proposito, questo scherzetto chi lo ha pagato? I compagni della Feltrinelli? Il genere letterario fantasma deve piacerle molto, però, perché vi state prostrando ai colossi farmaceutici con contratti segreti e tutti sbilanciati a favore di Big Pharma (lo stanno scrivendo un po' tutti, anche «L'Espresso» di questa settimana; l'«Huffington Post» titola: «Contratti segreti per i vaccini. L'Europa si arrende a Big Pharma»). Lo fa l'Europa? Beh, mica a caso. Lo fate fare a quell'istituzione che risponde alle multinazionali. A noi non interessa quante dosi state comprando: vogliamo vedere i contratti dalla prima all'ultima riga, senza restrizioni, perché siamo stati eletti dai cittadini italiani, non dai *manager* delle multinazionali. Provate a rendere obbligatorio il vaccino e a emettere patentini senza che questo Parlamento abbia visto i contratti d'acquisto dalla prima all'ultima riga: provateci, e vi promettiamo una resistenza che nemmeno ve la sognate. Non bisogna perdere la memoria, ha detto, ma a quale fate riferimento? A quella delle informazioni che state diramando con arbitrio menzognero? Quest'Assemblea deve conoscere il documento stilato da alcuni ricercatori indipendenti dell'OMS che il vostro compare Ranieri Guerra ha fatto togliere di mezzo, come ha chiaramente provato la trasmissione «Report». Per colpa del suo Ministero, l'Italia non aveva un piano pandemico, a meno che non vogliate prenderci in giro con i vari copia-incolla: per questo avete brigato con Ranieri Guerra, per impedire che i cittadini sapessero delle vostre mancanze. Non avete protetto gli italiani, anzi, avete violato il diritto costituzionale alla salute e poi, per proteggervi, avete tolto altre libertà e diritti costituzionali, dalla libertà di circolazione al diritto al lavoro e a fare impresa. Non solo: state intaccando anche il diritto a una giustizia autonoma, perché con il vostro silenzio state impedendo alla procura di Bergamo, che indaga per epidemia colposa, di interrogare il personale OMS scomodo. Lei e Di Maio avete ricevuto una lettera imbarazzante dall'OMS, che oppone l'immunità diplomatica per il suo personale (tutti, eccetto il solito Ranieri Guerra). Bonafede non ha niente da dire di tanta arroganza? Ranieri Guerra ha tutte queste coperture perché sta coprendo sé stesso, lei e il Governo sull'assenza del piano pandemico. Avete barattato le vite di 50.000 cittadini italiani in cambio del silenzio su un *dossier* che dice la verità sulle vostre colpe. Avete barattato le vite di 50.000 italiani in cambio di un video marchetta dell'OMS a cui avete appena dato un obolo di 10 milioni. Senza verità e senza trasparenza c'è solo la vostra propaganda. Basta segreti, basta menzogne: vogliamo la vera verità sui morti del Covid.

dopo l'altra tragica giornata del 18 novembre 2013, quando si verificò una situazione analoga a quella occorsa sabato scorso,

Tutti avete visto le immagini drammatiche di Bitti, dove l'acqua e il fango hanno superato il primo piano delle abitazioni e tre persone sono morte travolte dalla furia di acqua e detriti. A questo riguardo, voglio rivolgere un pensiero di cordoglio e vicinanza ai familiari delle persone decedute, a tutta la cittadinanza del Comune di Bitti e, in particolare, al sindaco Giuseppe Ciccolini: si tratta di un giovane sindaco, ottimo amministratore, a cui tutti dobbiamo un grazie sentito, perché, memore di quanto accaduto e sofferto nel 2013, aveva tempestivamente emanato in questa circostanza misure per mettere in sicurezza la cittadinanza, consentendo di limitare il numero dei morti soltanto a tre, che sono deceduti purtroppo per un'imprudenza da parte loro e solo per questo motivo; è un giovane sindaco che davvero ha saputo affrontare l'emergenza che si è venuta a creare in questa circostanza. Solidarietà dovuta e sentita sicuramente anche a tutti i Comuni colpiti dal nubifragio del 28 novembre, che non hanno dovuto dare un tributo di vite umane, ma sicuramente hanno avuto danni ingentissimi alla loro economia, con la distruzione di terreni e allevamenti andati distrutti. Mi riferisco in particolare ai tre Comuni che hanno avuto i danni più gravi (Galtellì, Onifai e Orosei). Adesso però dobbiamo evitare che la vicenda tragica finisca nel dimenticatoio, come troppo spesso è accaduto. Alle parole di cordoglio è necessario far seguire fatti concreti. Non posso non ricordare che oggi, dopo sette anni dalla vicenda del 18 novembre 2013, il ponte di Monte Pinu, che collega Olbia con Tempio Pausania, è ancora distrutto.

quella giornata tragica prestava servizio, proprio per questioni di sicurezza, al fine di cercare di contenere i danni alle vite umane. Quel ponte è stato sistemato soltanto l'anno scorso, dopo sei anni.

all'inizio della legislatura era stata istituita l'Unità di crisi Italia sicura; se ci fosse stata, probabilmente questo danno sarebbe stato evitato. Nonostante questo, il sindaco di cui ho già parlato si era dato da fare

Governo non valuti di dare un segnale forte e chiaro a una popolazione orgogliosa e fiera come quella di Bitti (chi non la conosce non può capire di cosa sto parlando), che non vuole l'aiuto dato tanto per darlo, ma qualcosa di concreto. Diamo un segno, per esempio, azzerando il debito tributario che in questo periodo

finestra"). La Presidenza, anche a nome dell'Assemblea, si associa nell'esprimere vicinanza e cordoglio alle famiglie colpite dal gravissimo lutto e solidarietà alla cittadinanza e a tutti i cittadini sardi.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, strade devastate, attività distrutte, famiglie rimaste senza una casa e vite spezzate: la Sardegna si è trovata di nuovo in ginocchio, davanti ad una bomba di acqua e fango che, con una forza mai vista negli ultimi decenni, ha lasciato tanta devastazione. L'ordine dei geologi ha sottolineato che questi nubifragi hanno evidenziato, ancora una volta, la fragilità dei centri urbani. Nonostante il susseguirsi di avvertimenti, si riscontra la mancanza di un'efficace politica di difesa del territorio incentrata sulla prevenzione del dissesto, attuabile con interventi finalizzati alla cura e alla disciplina del suolo. I centri rurali colpiti sono Bitti, Lula, Dorgali, Oliena, Nuoro, la valle del Cedrino, oltre a Torpè, Siniscola e Posada devastati dalle acque. Il settore agricolo fa la conta dei danni che, dai primi monitoraggi effettuati, risultano ingenti in molte parti della Sardegna. L'acqua ha inondato i campi dalla Baronia al basso oristanese, dal Medio Campidano al Sarrabus; in Ogliastra tantissime strade rurali e ponti distrutti hanno isolato gli ovili; molte aziende sono rimaste senza corrente elettrica e senza acqua, molti ettari di erbai dilavati e scorte di foraggio e mangimi bagnate. Nella zona di Villacidro, a San Gavino, Guspini e Gonnosfanadiga ci sono stati campi dilavati e l'allagamento di capannoni e fienili per via dello straripamento dei fiumi. È essenziale e di massima priorità agire con un piano di messa in sicurezza e di prevenzione nel territorio. Mi trovo d'accordo con il collega Cucca, ritenendo che è stata una mossa miope e pericolosa cancellare l'unità di missione «Italia sicura» senza sostituirla o applicando le dovute modifiche per renderla più performante. È fondamentale salvaguardare le aree a rischio idrogeologico e realizzare concrete missioni per la lotta al dissesto.

adesso quello agricolo, che rimaneva una forte speranza per trainare l'economia sarda. La procedura per richiedere lo stato di calamità al Governo è stata avviata; il presidente Solinas ha stanziato 40 milioni di euro per un ristoro immediato a favore delle comunità maggiormente colpite dalla furia del ciclone *(Applausi);* Confagricoltura richiede l'utilizzo del *recovery fund* a sostegno del settore agricolo. Personalmente ringrazio di cuore le forze dell'ordine, la Protezione civile, le centinaia di volontari intervenuti immediatamente sui luoghi. È con immenso cordoglio che esprimo la mia solidarietà a tutti i miei conterranei, vittime di questa tragedia. Tuttavia, come scriveva il nostro premio Nobel Grazia Deledda, nel romanzo «Canne al vento», il rimedio è in noi e sono certa che il popolo sardo si dimostrerà resiliente e si rialzerà con la forza e la determinazione di sempre. *(Applausi)*.

devastazione che si è prodotta a seguito del maltempo di sabato scorso, 28 novembre, per cui oggi siamo al secondo giorno di lutto cittadino. Come Forza Italia tengo a rappresentare la partecipazione al cordoglio dei familiari. Come politico intendo sottoscrivere ciò che hanno proposto i colleghi Lunesu Lunesu e Cucca riguardo allo stato di calamità naturale ed un intervento che sia risolutivo rispetto ai danni già prodotti circa sette anni fa nella stessa zona. Sono sicuro che presidente Solinas, in accordo con il Governo, troverà le soluzioni migliori affinché non si debba tornare altre volte a piangere i lutti e a riparare i danni che l'ambiente sempre di più sta subendo in zone devastate come quella di Bitti.

Il fiume che attraversa il paese, raccolto in un canale tombato oramai vetusto, a causa di una bomba d'acqua violentissima è uscito dal suo letto e ha attraversato la via principale del paese con una furia incontrollabile, quattro volte maggiore di quella che si era vista con il ciclone Cleopatra nel 2013. Ai bittesi, popolo mite e semplice di grandi lavoratori, va tutto il mio cordoglio in questo momento così drammatico. Con molta dignità loro stessi, aiutati in questi giorni dalle Forze dell'ordine, dall'Esercito, dai Vigili del fuoco, dal Corpo forestale cui va tutto il mio ringraziamento, stanno lavorando per liberare il paese dagli enormi mucchi di detriti e di fango. Non ho sentito da parte loro alcuna rabbia o alcuna ricerca di responsabilità, alcun puntare il dito, ma come cittadina, prima ancora che come una responsabilità la sento addosso, perché ancora una volta ci siamo fidati di infrastrutture obsolete. Poco è stato fatto dal 2013 ad oggi per mettere in sicurezza il paese sotto il profilo del contenimento e quindi del rimboschimento e sono mancati anche le necessarie importanti opere idrauliche. Ormai il cambiamento climatico accelera questi eventi, che infatti sono sempre più frequenti, ma evidentemente il piano idrogeologico regionale, che individua le aree caratterizzate dal più alto rischio, non ha trovato in questi anni adeguata applicazione. Spesso si fanno progetti e si mettono in campo finanziamenti, ma poi il tempo passa, senza che nulla di fatto accada. L'eccessiva burocrazia blocca tutto, ma anche il famigerato consenso della politica. Gli amministratori locali devono imparare a dire di no; non è più pensabile costruire sul letto dei fiumi. Occorre impedire ai cittadini un uso distorto del territorio che metta in pericolo la loro stessa vita. vita. Presidente, concludo allora auspicando che il Governo stia vicino alla mia comunità, quella di Bitti, con tutto il supporto necessario e finanziario per la ricostruzione del Paese e la messa in sicurezza del territorio. Mi unisco all'appello dei miei colleghi sardi, affinché la comunità sia aiutata anche con un azzeramento della tassazione e sia naturalmente dichiarato lo stato di calamità naturale. Ringrazio l'Assemblea

Stavolta c'è stato detto che andava fatto a fine seduta e ora lo facciamo a fine della fine seduta, quando i nostri colleghi parlamentari hanno lasciato quest'Aula.

Lo faccio leggendo quello che un autorevole giornalista ha scritto proprio in merito al deserto - morale, prima ancora che politico - di quest'Aula. Lo ha fatto due giorni fa sul «Corriere della Sera» Pierluigi Battista, scrivendo dei 18 pescatori dimenticati in Libia, e il fatto che ne debba parlare in un'Aula deserta, ovviamente nell'assenza del Governo, è emblematico di quello che già lui ha scritto in questo articolo che vi leggo:

Insomma sono ostaggi, catturati e usati come merce di scambio con l'Italia. Ma l'Italia non ha alcuna intenzione non dico di scambiare alcunché, ma di prendere in considerazione l'idea stessa di una trattativa per liberare diciotto nostri connazionali nelle grinfie di bande armate cui è difficile riconoscere dignità statale. Colpa di un Governo palesemente inadeguato come quello italiano, certamente, senza una *leadership*, un minimo di peso internazionale, uno straccio di profilo che possa incutere rispetto. Ma colpa anche di un'opinione pubblica silente, indifferente, messa a tacere da un misto di fatalismo, di disattenzione, di assuefazione» (parlo, appunto, in un'Aula deserta, disattenta, assuefatta). «E c'è davvero da domandarsi perché. Perché la sorte di diciotto pescatori non ci muova a un minimo di solidarietà. Guardiamo la notizia, non ne veniamo toccati, la prendiamo come una noiosa incombenza. Siamo gonfi di indignazione, di vibrante protesta per la scandalosa detenzione in Egitto dello studente Patrick Zaki, conosciuto all'Università di Bologna, e facciamo bene a protestare, a firmare appelli, a richiamare l'attenzione su questo sopruso. Ma perché niente, il nulla assoluto, il mutismo illimitato sui diciotto pescatori. Facciamo sentire il nostro plauso quando qualche cooperante, o qualche giornalista, viene liberato dopo lunghe e onerose trattative, ma del destino di diciotto pescatori sequestrati non ci importa niente, come se l'umanità di diciotto sconosciuti non ci riguardasse (...) o fosse meno "di tendenza" occuparsene, protestare, chiedere la loro liberazione». «E questa volta nemmeno l'opposizione di destra, un tempo combattiva e indignata per i due marò prigionieri in India, sembra commuoversi. Come se fossero italiani di un'Italia minore, appartenenti a una categoria troppo umile» (i pescatori) «per alimentare la nostra coscienza morale incostante, spaventosamente ipocrita, di un'ipocrisia così incistata nel nostro modo strabico di vedere le cose che forse nemmeno riusciamo a rendercene conto. Perché i Perché i pescatori non contano niente, non fanno opinione, non invitano alla mobilitazione. E se ne stanno lì, sotto sequestro da novanta giorni, nel silenzio del mondo». E aggiungo, nel silenzio di un'Aula deserta come questo Senato della Repubblica. Grazie,

intervenire a fine seduta in un'Aula praticamente deserta - ringrazio i pochi colleghi rimasti - è anche difficile; sembra quasi oltraggioso per chi è costretto a rimanere qui ad ascoltare, quindi cercherò di essere assolutamente breve.

898 del 1970 istitutiva del divorzio, ovvero la legge Fortuna-Baslini. Intervengo anche in quanto senatore del Friuli-Venezia Giulia, essendo Fortuna un friulano, o meglio un lombardo che in tenerissima età si è trasferito a Udine: il papà era cancelliere del tribunale di Udine, poi lui divenne avvocato penalista,

deputato. Uno dei suoi primi atti più importanti fu quello di presentare una proposta di legge sull'istituzione del divorzio, sulla scia di quanto

cui in Italia e in Europa c'era il terrorismo e, nonostante tutto, il Parlamento, pur nelle divisioni ideologiche profondissime che lo contraddistinguevano tra le varie forze, riusciva a produrre queste leggi.

di molte persone, compresi anche coloro che, per motivi ideologici, contrastavano questo fronte: penso alla Democrazia cristiana di Fanfani

i cosiddetti sentimenti sono cangianti e deboli e quindi, di conseguenza, il tema del vincolo e della sua indissolubilità non poteva essere sottratto a ciò che contraddistingue l'essere umano e quindi anche alla mutevolezza dei suoi sentimenti.

Grazie,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei parlare del lunghissimo viaggio della speranza che ha condotto a Napoli, proveniente dal Venezuela, un bimbo di sei anni che, accompagnato dai propri genitori, si è affidato ai medici specialisti napoletani con una profonda speranza nel cuore e una grande voglia di vivere. Il suo fisico, esile, gracile e stremato dalla malattia oramai sembrava essere sopraffatto dalla forma grave di leucemia linfoblastica acuta che l'aveva colpito, aggravata dalla concomitante presenza del virus dell'epatite C, contratto quest'ultimo nel corso delle terapie e delle trasfusioni praticate nel suo Paese originario. Gli ematologi dell'ospedale Santobono Pausilipon hanno eseguito un trapianto di cellule staminali del midollo osseo, ottenendo una buona risposta terapeutica da parte del piccolo e una remissione della sua malattia ematologica. Il lavoro, coordinato col centro di patologia dell'Università Federico II di Napoli ha permesso di superare anche le barriere burocratiche che vietavano, fino a poco tempo fa, l'utilizzo al di sotto dei dodici anni di età dei nuovi farmaci antivirali per sconfiggere l'epatite C. Dopo circa tre mesi di cure secondo i protocolli terapeutici internazionali, il midollo del piccolo è guarito o, come si dice in termine medico, è pulito e al tempo stesso il virus dell'epatite C si è negativizzato. Presto il piccolo potrà ritornare in Venezuela. In un momento storico così particolare questo episodio rappresenta un messaggio positivo per tutti noi e dimostra ancora una volta che le competenze e le professionalità dei nostri medici e dei nostri operatori sanitari sono unite sempre ad umanità, sensibilità e disponibilità anche nell'accogliere bambini provenienti da Paesi lontani, con una richiesta di aiuto e una mano tesa che va oltre i confini territoriali. È bello pensare che nella mia Campania, regione così devastata dalla pandemia, possa nascere e diffondersi un messaggio di speranza nel futuro, in uno spirito di solidarietà e di vicinanza tra persone di Paesi e di continenti diversi.

mi rivolgo al Parlamento affinché solleciti il Governo ad attivarsi sulla vicenda dello scienziato iraniano-svedese Ahmad Jalali, imprigionato dal Governo iraniano nel 2016. Era stato invitato a tornare nella sua nazione di nascita per una conferenza ed è stato arrestato con l'accusa di spionaggio condannato a morte nel 2017. A quanto si apprende in questi giorni da Iran human rights, potrebbe essere giustiziato oggi stesso o nei prossimi giorni. Ahmad è un medico che si occupa di medicina dei disastri, è cittadino svedese e cittadino europeo, oltre che iraniano, ha svolto le sue ricerche in Svezia e in Belgio, ma anche per un lungo periodo in Italia presso l'Università del Piemonte orientale di Novara e, pur avendo proclamato la sua innocenza rispetto alle accuse di spionaggio, oggi davvero rischia la vita la vita a causa dell'*escalation* di tensioni geopolitiche molto più grandi di lui. È ovvio anche che la sua storia e l'accusa che gli viene mossa non può non farci ricordare la tragedia e la triste storia di Giulio Regeni, per il quale non abbiamo potuto fare nulla perché abbiamo saputo troppo tardi. Per Ahmad, invece, sappiamo dov'è e sappiamo che oggi è vivo. Come cittadini dell'Europa, spazio di libertà e democrazia di riferimento per tutto il mondo, non possiamo permettere che un uomo, un padre, uno studioso venga giustiziato senza la possibilità di un giusto processo, sulla base di accuse che ha sempre negato. Chiedo dunque al Parlamento che si appelli al Governo, in particolare al presidente del Consiglio Conte e al ministro degli affari esteri Di Maio, affinché prenda in considerazione ogni iniziativa volta a sospendere la partecipazione del nostro Paese ad accordi che facilitano l'interscambio accademico tra Italia e Iran, attivandosi, insieme alle massime autorità europee, per ottenere la sospensione di ogni procedimento giudiziario che possa portare alla morte di Ahmad Jalali e ripristinare la garanzia che la sua detenzione rispetti il diritto internazionale. La condanna a morte di un ricercatore, di chi non coltiva altro che la conoscenza, credo debba essere vissuta dalla comunità internazionale come un attacco portato al cuore del nostro modello di convivenza, al pari di un'aggressione al corpo diplomatico o ad un soldato in servizio di *peacekeeping.*

accordi e come preannunciato, sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, che è stata convocata per le ore 15 fino alle ore 16. La seduta è sospesa.

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 18 dicembre. L'Assemblea si riunirà mercoledì 9 dicembre, alle ore 16, per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020. Nella settimana successiva, con sedute da lunedì 14 dicembre, alle ore 16,30, fino a venerdì 18, se necessario, saranno discussi il decreto-legge ristori e il decreto-legge immigrazione, quest'ultimo attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. Il calendario potrà essere integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato. In relazione alle determinazioni limitative riguardo alla programmazione dei lavori delle Commissioni nell'attuale fase di emergenza i Capigruppo hanno convenuto di autorizzare la Commissione giustizia a proseguire l'esame, in sede deliberante, del disegno di legge concernente la proroga della Commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti